Signor Presidente, il decreto-legge in esame, nel testo approvato alla Camera dei deputati, contiene misure urgenti per il settore energetico. Il testo originariamente trasmesso al Parlamento era composto da quattro articoli, ma le disposizioni contenute nei primi due, relative a misure per gli enti territoriali e per la tempestiva attuazione del PNRR, sono state successivamente trasfuse nel decreto-legge n. 51 del 2023, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 28 giugno. Conseguentemente, tali articoli sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del suddetto decreto-legge n. 51. Durante l'esame alla Camera dei deputati, nel provvedimento in esame è stato poi riversato il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, relativo a misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ovvero l'ultimo decreto bollette. Tale articolo è dunque abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione in esame e il suo contenuto è riprodotto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge. L'8a Commissione del Senato non ha apportato modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, ma durante l'esame sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno, in larga parte delle forze di opposizione. Venendo al contenuto degli articoli del decreto-legge, come si è detto, gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dalla citata legge n. 87 del 2023. L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale,

*relatrice*. In particolare, il comma 1 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze di autorizzazione ai commissari straordinari di Governo già nominati. Il comma 2 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le autorizzazioni vengano rilasciate dal competente commissario straordinario a seguito di un procedimento unico, della durata massima di 200 giorni, che comprende anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre la disciplina precedente aveva previsto un termine di centoventi giorni e l'esenzione delle valutazioni ambientali. Il comma 3 apporta una serie di modifiche testuali al suddetto articolo 5 del decreto-legge n. 50. In particolare, la lettera *a)* precisa che la finalità della nomina dei Commissari straordinari non è solo la realizzazione, bensì la realizzazione ovvero l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture per l'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete. La novella al comma 5, introdotta dalla lettera *b)*, stabilisce conseguentemente che le istanze ai Commissari straordinari possano essere presentate non solo dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, ma dai soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle stesse. La lettera *b-bis)* impone ai Commissari straordinari di provvedere tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina il diritto di accesso nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con la lettera *c)* si interviene sul comma 14-*bis*, precisando che la disciplina sulle unità galleggianti ivi contenuta si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, di dette unità, rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. La lettera *d)* introduce il nuovo comma 14-*ter*, ai sensi del quale, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti. Il comma 4 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), con conseguente applicazione ad esse della disciplina speciale che riguarda tali progetti. Come è stato anticipato, l'articolo 3-*bis* recepisce il contenuto dell'ultimo decreto bollette. In particolare, il comma 1 prevede che, per il terzo trimestre del 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro

Il comma 4 proroga, sempre per lo stesso periodo dell'anno, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali. In base al comma 5, tale agevolazione è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. I commi 3 e 6 recano le disposizioni per la copertura

in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi I criteri per la definizione dei prezzi minimi garantiti e delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico prevedono che tali agevolazioni - il cui valore deve essere aggiornato annualmente siano corrisposte a copertura dei costi di funzionamento degli impianti e siano differenziate in base alla potenza di questi ultimi. Gli impianti inoltre devono rispettare i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021. L'articolo 3-*quater* integra l'articolo 1 del decreto-legislativo n. 22 del 2010 in materia di coltivazione delle risorse geotermiche. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che i soggetti titolari di permessi di ricerca finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza (trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento) nell'ambito della successiva richiesta di concessione possano presentare contestualmente istanza di potenziamento, con una variazione del programma dei lavori. In tal caso, non si applicano i limiti di potenza nominale installata e di energia immessa nel sistema elettrico, previsti dalla normativa vigente. L'articolo 3-*quinquies* modifica il regime autorizzatorio applicabile agli impianti di produzione di biometano. In particolare, il comma 1 stabilisce che siano sempre sottoposti a procedura abilitativa semplificata gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica inoltre le condizioni al sussistere delle quali possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica, gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione. Il comma 2 estende le agevolazioni sulle accise previste dalla normativa vigente per il gasolio commerciale anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio. L'articolo 3-*sexies* introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico. In particolare, il comma 1, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, qualifica come infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione, ovvero il cui efficientamento, siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord, ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei. Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni attribuiscono priorità ed urgenza alle procedure autorizzative nelle quali esse siano a qualunque titolo coinvolte. Ai sensi del comma 2, per la realizzazione e l'efficientamento delle infrastrutture energetiche strategiche, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità,

articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con

le attività finalizzate alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo svolte dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali. L'articolo 3-*octies* prevede che, per le procedure d'asta indette dal GSE per l'assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella normativa vigente - e in particolare nel decreto ministeriale 4 luglio 2019 - siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del

Presidente, colleghi, penso che la discussione di oggi sia un altro tassello della nostra riflessione sul tema del PNRR, un tassello che si aggiunge agli svariati tentativi di questo Governo cambiare approccio su alcune questioni, anche modificando atteggiamento sul tema dell'energia nella direzione giusta, perché non c'è dubbio che rispetto agli impianti, alle posizioni molto timide che questa destra che governa ha avuto in passato, addirittura ostili rispetto alla necessità di trasformare e di modernizzare il Paese, c'è stata una virata una virata consistente, una di quelle virate nelle quali voi siete esperti, campioni mondiali di ribaltamento di impostazione, vi siete ritrovati da un approccio populista e demagogico a dover fare i conti con la realtà della vita e delle cose, con l'aumento del costo dell'energia e con le difficoltà che gli italiani hanno hanno vissuto. Avete così riscoperto il realismo, ma - intendiamoci - noi siamo sempre molto contenti quando percepiamo una trasformazione di atteggiamento rispetto a posizioni che invece Italia Viva ha sempre tenuto con coerenza, anche quando le proteste erano violente, anche quando non c'era da guadagnarci facili consensi, anche quando era difficile affrontare questi temi con l'opinione pubblica. Ma noi siamo fatti così, siamo gente testarda convinti che la coerenza alla fine paghi, non so se dal punto di vista elettorale, ma sicuramente rispetto alla nostra dignità di forza politica che crede nel cambiamento e che ha fiducia nel Paese. da parte di questo Governo, un cambiamento radicale di impostazione. Oggi credete nel rigassificatore, a Piombino avete tenuto un atteggiamento ambiguo,

con le conferenze dei servizi che non terminano mai, con una burocrazia che non consente di far fare passi in avanti sui temi che sono importanti anche per renderci maggiormente autonomi dal punto di vista energetico, ma anche per strutturare un Paese che ha una vocazione industriale e produttiva di tutto rispetto. All'interno di questo decreto ci sono, obiettivamente, delle semplificazioni che vanno in quella direzione. E allora perché il nostro è un atteggiamento critico? È critico perché non dobbiamo dimenticarci che intanto voi affrontate questa discussione, che sarebbe del tutto naturale fare con un ragionamento d'Aula privo di forzature, all'interno di un voto di fiducia. Quindi compromettete questa discussione dal punto di vista del merito, perché la sommate a valutazioni politiche che ovviamente ci rendono impossibile addentrarci nelle singole questioni. Però non voglio fare di questo il vero discrimine rispetto alle nostre critiche, perché le nostre critiche sono di natura più generale.

Ha provato invece a instaurare un dialogo con le Aule parlamentari. Ma veniamo alla sostanza: ci sono davvero dei passi in avanti sulla questione del PNRR che possono essere apprezzati? Questo è il tema. Vi do un'informazione: giratevi il Paese, perché di opere che stanno partendo sul PNRR io ne vedo pochissime. Voi potete anche continuare a raccontare quella dell'uva e delle responsabilità di quelli che c'erano prima; ma al Governo ci siete voi da otto mesi. Continuiamo a parlare di cabina di regia, continuiamo a parlare di modificare un progetto rispetto all'altro, continuiamo a dire che Draghi forse non aveva fatto il PNRR migliore di questo mondo. Io accetto tutto, anche le critiche più spietate. Ma, dopo otto mesi, ci volete dire quali progetti non partono e quali progetti intendete attuare? Questo è il tema

con la mano sinistra, non si chiarisce quali sono le priorità reali del Paese, quali sono i rigassificatori che si vogliono costruire, quali sono i dissalatori che si vogliono realizzare, quali sono le opere infrastrutturali che si vogliono mettere in campo. Parallelamente a questo, si vende un processo di semplificazione, come per esempio il codice degli appalti, come la panacea di tutti i mali. Anche qui vi do un'informazione: voi ci batterete con il naso su questa questione, perché alla fine è quello che non partirà a dare il giudizio sull'operato di questo Governo, che può raccontare di un condono un giorno, di un di un reato il giorno successivo, ma alla fine sarà giudicato per quello che sarà in grado di realizzare. Vi do una notizia: il codice degli appalti voluto da Salvini non è affatto in grado di semplificare, anche perché c'è un problema a monte, nell'*iter* autorizzativo e nella fase progettuale, che vi guardate bene dal mettere in campo e dal migliorare. Quindi, da un lato, si introducono principi anche corretti; dall'altro, però, non si ha un'azione organica di semplificazione, ma un tentativo maldestro di mettere toppe qua e là. Poi c'è un tema, che io penso sia giusto ribadire in questo contesto. Dentro questo decreto intervenite nuovamente sulla questione delle bollette. Benissimo, ogni euro che gli italiani risparmiano è un fatto positivo. la rideterminazione delle tariffe la modulate nel limite di 110 milioni. Beh, amici, siamo ben lontani dai crediti di imposta, dalle detrazioni, dalla strategia Draghi su questo tema. La coperta è corta, lo capiamo perfettamente; però voi avevate iniziato questo percorso di Governo nel Paese dicendo che vi sareste occupati delle accise sulla benzina, ma non c'è stato un intervento strutturale, nonostante la modificazione dei costi dell'energia, che rende ingiustificabile quello che gli italiani stanno pagando in termini di aumento dei costi sulla benzina. Parallelamente, state restringendo il perimetro della strategia di aiuto alle famiglie in un momento di massima difficoltà.

per fare un intervento incisivo sul credito d'imposta; ma utilizziamo queste risorse anche per contrastare i rincari, che sono una spada di Damocle sulla testa delle famiglie italiane. Questo è quello che voi avreste dovuto fare dovuto fare e che avreste dovuto scrivere in questo decreto-legge di rimodulazione del PNRR. Vi aspettiamo al varco della discussione della prossima settimana, con il ministro Fitto, quando dovrete cominciare a dire quali sono i progetti. Vi do un'altra informazione. Mentre parliamo di opere sostitutive, state rimodulando i contratti di programma di RFI tagliando tante opere ferroviarie perché non siete in grado di farle partire. *(Applausi)*. Altro che Paese che si muove: lo vediamo in questi giorni cosa sta succedendo con i treni e con il caos nel Paese. Il gesto di debolezza che fate oggi, cioè apporre la fiducia su un decreto-legge tutto sommato semplice, la dice lunga sull'incapacità e sulle difficoltà che per i mesi di ottobre inizio a vedere molto serie per questa maggioranza, ed è la ragione per la quale ci ritroveremo qui senza farvi sconti; senza alcun alcun atteggiamento ideologico, ma nemmeno accettando il fatto che, dopo aver raccontato che avreste cambiato l'Italia, la state immobilizzando ad un destino assolutamente incerto.

ai dati economici, ai dati Istat e di organismi terzi che dicono tutt'altro rispetto a quanto oggi sentito in Aula dalla collega Paita. *(Applausi)*. Il Paese reale che organismi terzi ci trasmettono e oggi ci restituiscono dice tutt'altro rispetto alle parole sentite sentite poc'anzi in quest'Aula. Veniamo al decreto-legge in conversione, che riguarda un settore che in momenti di normalità per qualsiasi Paese sarebbe strategico. Immaginiamo quello che invece è e può essere oggi,

russo-ucraina si sono mostrate tutte queste fragilità e siamo dovuti intervenire, anche perché gli approvvigionamenti non sono più arrivati. Ci siamo resi conto di un problema che conoscevamo e lo abbiamo affrontato; quindi oggi e in questi anni, anche come Forza Italia e come centrodestra, stiamo risolvendo questo problema. Un grande lavoro è stato fatto e tanta strada è stata percorsa.

otto mesi è dovuto intervenire in molte situazioni che riguardano sia il PNRR, per la cosiddetta messa a terra, sia oggi le politiche energetiche. Questo è quindi il quadro che andiamo oggi a rivedere. Si rende dunque necessaria una revisione delle nostre politiche energetiche, anche perché dobbiamo guardare in un quadro internazionale mutato e difficile e soprattutto perché, come dicevo, è un punto centrale

cercare di essere come Paese quanto più autonomi nella produzione di energia. Cambiano dunque alcune regole, soprattutto per quanto riguarda le unità galleggianti di stoccaggio e di rigassificazione; abbiamo l'estensione da centotrenta a duecento giorni (quindi fino al 29 luglio del 2023) del procedimento autorizzativo di rilascio di queste autorizzazioni, comprensive anche di valutazione di impatto ambientale.

dell'importo sulle bollette per quanto riguarda il gas metano per gli usi civili e combustioni industriali, sia per il mese di luglio che per i mesi di agosto e di settembre 2023. decreto sono 285 milioni di euro che mettiamo oggi a sostegno delle famiglie e delle nostre imprese per quanto riguarda l'energia elettrica. Se a questo ci aggiungiamo

della grande crisi che abbiamo vissuto in questi anni - a circa 30 miliardi di sostegno e di aiuto diretto alle famiglie e alle imprese per sostenere i costi dell'energia elettrica, pari all'1,3 per cento del PIL: l'intervento dell'Italia

con un emendamento che è stato presentato e approvato, concerne una procedura abilitativa semplificata proprio per le riconversioni alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione. Quindi, questa è un'ulteriore fonte di approvvigionamento che noi mettiamo

a queste fonti: quindi, si riprende quello che era stato scritto già nel decreto-legge n. 50 del 2022 all'articolo 5, dove si definivano i rigassificatori galleggianti come degli interventi strategici di pubblica utilità indifferibili. Quindi, l'articolo 3 riprende un articolo del precedente decreto e così diamo seguito anche all'utilizzo dei rigassificatori Non abbiamo, dunque, grandi novità su questo decreto, ma vi confermiamo la politica di sostegno ed aiuto alle imprese con ulteriori risorse; continuiamo sulla strada della semplificazione delle autorizzazioni per quanto riguarda altri impianti e quindi la produzione di energia. Con coerenza, dunque, noi di Forza Italia e il centrodestra andiamo avanti su questa strada.

Vengo ora all'impegno del Ministro di Forza Italia, il ministro Pichetto Fratin, che in questi mesi si sta impegnando tantissimo su questo tema. esame riesca a contemperare con equilibrio il ricorso alle fonti di produzione consuete, quelle che conosciamo tutti, con il ricorso a fonti alternative e con l'incentivazione e la semplificazione della diffusione di energie rinnovabili.

del Governo, davanti a questo ennesimo decreto farsa, vorrei provare a fare un ragionamento un po' più ampio. Sono nove mesi che questo Governo continua ad emanare provvedimenti bandiera che non risolvono in alcun modo le difficoltà dei cittadini, anche provvedimenti sbagliati. E sono sbagliati, perché non tengono conto del contesto nazionale, del contesto europeo e del contesto internazionale Se questa maggioranza e questo Governo non l'hanno capito, oggi il vero problema sono le disuguaglianze, che sono le più ampie di sempre. Nei giorni scorsi è stata pubblicata un'accorata lettera, firmata da 236 economisti ed intellettuali provenienti da 67 Paesi. questa lettera, firmata da nomi come Joseph Stiglitz e Mariana Mazzuccato ed indirizzata alle Nazioni Unite ed alla Banca mondiale, questi intellettuali ed economisti

mentre la metà più povera della popolazione guadagna l'8,5 per cento. Quindi, si chiedono nuove forme di monitoraggio e di potenziamento dell'obiettivo delle Nazioni Unite di riduzione delle disuguaglianze. Invece, colleghi, tutti i provvedimenti di questo Governo non fanno altro che andare nella direzione opposta. Farò qualche esempio: la delega fiscale polverizza il sistema fiscale in tante *flat tax* che contrastano con l'equità orizzontale e verticale, come denunciato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti e dalla Banca d'Italia. Il decreto-legge, che voi chiamate lavoro e noi chiamiamo precariato, non fa altro che precarizzare e impoverire ancora di più i lavoratori. Per non parlare delle parole del ministro Tajani sul salario minimo: sono parole che fanno venire i brividi, signor Presidente, perché richiamano, a mio avviso, quella corrosione del linguaggio che l'economista francese Fitoussi, riprendendo Orwell, definiva neolingua, cioè un linguaggio creato ad arte per limitare la comprensione dei cittadini. signor Presidente, la neolingua della nostra epoca è, ad esempio, far credere che a vivere di rendita non sono i grandi colossi finanziari, ma i poveri che hanno osato chiedere protezione sociale, i disoccupati, i lavoratori poveri. La neolingua del ministro Tajani fa credere che col salario minimo si vogliano impoverire anche tutti gli altri lavoratori, quando invece è esattamente l'opposto. Del resto, in nessuno dei Paesi europei in cui il salario minimo è stato già introdotto c'è stata una diminuzione dei salari. signor Presidente, piace invece la lingua della Costituzione, che all'articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a se stesso e alla propria famiglia. Parlando ancora dei provvedimenti della maggioranza, che non faranno altro che aumentare le disuguaglianze, voglio fare un cenno all'autonomia differenziata, un progetto scellerato che provate

A fronte di questi provvedimenti che aumentano le disuguaglianze, non riuscite nemmeno ad utilizzare le risorse di quell'unico strumento che abbiamo oggi per eliminare le disuguaglianze, che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Signor Presidente, qui c'è un dato di fatto e anche in questo caso basta guardare i numeri. Dei 33 miliardi di euro previsti per la spesa del nel 2023, ad oggi sono stati spesi solo 2 miliardi di euro, nonostante la terza e la quarta rata siano già inseriti nel bilancio dello Stato. Davanti alle parole del ministro Fitto, che prova a spargere tranquillità, in realtà vorremmo fare solo due semplici domande: come pensa il Ministro, in questi sei mesi, di spendere i 30 miliardi di euro che non sono stati spesi

avete aumentato le disuguaglianze anche con la legge di bilancio e con il DEF che avete approvato, in cui avete seguito un'unica ricetta, quella dell'austerità, che si è tradotta in tagli alla spesa pubblica

tagli al reddito di cittadinanza, tagli ad opzione donna, tagli alle rivalutazioni delle pensioni medie, ai fondi per affitti e morosità incolpevole, tagli ai *bonus* edilizi e alla transizione 4.0. Infatti, al senatore Damiani, che prima parlava di andare a rivedere i dati, vorrei dire di andare a rivedere i dati del

Insomma, solo tagli ed è preoccupante, perché invece dovremmo andare a ridurre le disuguaglianze. Vediamo invece che anche nella delega fiscale che avete appena approvato alla Camera dei deputati non c'è un euro per ridurre le tasse, perché è a invarianza di gettito. Del resto, come pensate di recuperare risorse se non avete il coraggio di andare a prendere quelle risorse lì dove ci sono, dagli extraprofitti dei colossi energetici e del settore bancario? Non ci saranno mai i soldi per diminuire le tasse a lavoratori e imprese se non avete il coraggio di andarli a recuperare. Del resto, noi questo centrodestra lo conosciamo, perché è lo stesso da vent'anni, che propone sempre le stesse ricette, mentre lì fuori, Presidente, il mondo oggi è incredibilmente cambiato. Passo brevemente a questo decreto farsa che discutiamo oggi, che dovrebbe contenere misure urgenti per il settore energetico, ma di misure non ce n'è neppure l'ombra, perché non c'è nulla per ridurre il costo delle bollette e non c'è nulla per portare il nostro Paese nella direzione dell'indipendenza energetica. Questo decreto-legge contiene pochissime misure e sono tutte pericolose, a nostro avviso, per il Paese. La prima misura è la riapertura dei termini per autorizzare, realizzare o ricollocare nuovi rigassificatori, individuando aree, come quella per esempio di Piombino, che è un'area di crisi complessa dal punto di vista industriale, sanitario e turistico; un'area che ha già dato tanto e non ha bisogno certamente di un rigassificatore. La seconda misura è quella che semplifica le procedure per espropriare i terreni dove si vogliono far passare gasdotti e oleodotti; insomma, si preparano affari per pochi e questi affari andranno invece sulle spalle di tutti i cittadini, perché il vostro piano Mattei, quello che volete rilanciare come piano energetico per l'Italia, in realtà non fa altro che candidare il nostro Paese a diventare uno snodo di tubi che vengono da altri Paesi. Passiamo semplicemente da un fornitore all'altro; il fornitore prima era la Russia, adesso è il Nord Africa, ma non andiamo nella direzione dell'indipendenza. Per raggiungere quella direzione tutti gli indicatori ci dicono Per raggiungere quella direzione tutti gli indicatori ci dicono che dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili. Invece voi continuate a spendere decine di miliardi di euro per i sussidi ambientalmente dannosi e ignorate tutti gli appelli che vi vengono fatti. Ignorate anche l'appello a limitare la decretazione d'urgenza entro i limiti costituzionali. Del resto, voi ignorate tutto ciò che non è funzionale ai vostri interessi e quindi ignorate i poveri, ignorate le liste d'attesa in sanità, ignorate la necessità di assumere nuovo personale sanitario, ignorate i costi delle bollette, l'appello degli enti locali ad essere coinvolti di più nella spesa dei fondi PNRR, ignorate i lavoratori poveri e sottopagati, ignorate evidentemente - lo leggiamo anche in questo decreto - l'emergenza climatica. Questo l'abbiamo percepito in maniera netta anche ieri in quella discussione surreale sul disegno di legge in materia di carne coltivata, dove una parte della maggioranza addirittura ha parlato di orticaria verso il *green*, ha detto che si usa il pretesto del cambiamento climatico e che la CO2 tutto sommato ha anche effetti positivi. io non credo che il Paese meriti di ascoltare in quest'Aula posizioni antiscientifiche, negazioniste e pericolose.

a dover discutere oggi in quest'Aula. Voglio concludere con un proverbio dei nativi americani, che diceva che quando avrete abbattuto l'ultimo albero, pescato l'ultimo pesce, inquinato l'ultimo fiume, solo allora vi accorgerete forse che il denaro non si può mangiare.

possiamo apprezzare un contenuto sempre di natura emergenziale che non si disgiunge da un'attenzione verso le categorie più deboli, che ancora oggi avere difficoltà a sostenere l'aumento del costo dell'energia che molte famiglie si vedono ancora addebitare nelle fatturazioni dalle società di fornitura.

delle nostre relazioni internazionali che stanno riportando l'Italia al centro di una visibilità per quanto riguarda la soluzione di problemi che ci hanno riguardato. Parlo anche del MoVimento 5 Stelle che in parte, nello scorcio dell'ultima legislatura, ha dovuto gestire questi problemi. La strategia di cui vorrei parlarvi è quella di aver finalmente risolto in pochissimo tempo un legame, che devo

per essere divenute teatro di grandi battaglie, come Dunkerque o Stalingrado. Io vengo dalla provincia di Livorno e se questa battaglia l'abbiamo vinta lo dobbiamo anche alla città di Piombino,

alle legittime reazioni della popolazione per il fatto di dover sopportare anche un carico ulteriore in termini di gravami ambientali,

la condotta *pipeline*; in un certo momento, quando Gazprom non poteva garantire il pagamento dell'affitto di quel passaggio, quel Paese ha bloccato il transito del gas, bloccando le forniture che il nostro Paese aveva già acquistato. Devo dire che con lungimiranza siamo riusciti, con un'azione diplomatica, a sbloccare quella fornitura di gas che si era interrotta. Questo è il motivo per cui il Governo oggi ritiene indispensabile considerare una strategia geografica del nostro Paese non egoisticamente valevole solo per l'Italia, ma per tutto il Continente europeo senso, all'azione del *premier* e di tutto il Governo nel momento in cui considera la possibilità di creare una sorta di *hub* nazionale e quindi anche una capacità infrastrutturale per trasmettere

non dobbiamo considerare questo un punto d'arrivo. Spero che non rimarremo dipendenti esclusivamente dal gas naturale liquefatto (GNL) e da altre fonti esclusive di fornitura strategica, che vedremo presto una diversificazione che tenga conto anche dell'energia nucleare, della capacità quindi di poter ripresentare al popolo italiano, attraverso tecnologie innovative, la possibilità di sfruttare anche una fonte di energia che può garantire stabilità per lo meno al settore energivoro industriale, che oggi è alle prese con particolari difficoltà nel far fronte a quei picchi di costi che non possiamo escludere si ripresentino, dato che il mercato è - ahimè - in qualche modo sottoposto alle mutevoli situazioni geopolitiche internazionali.

è finalizzata soltanto a valutare le singole azioni di dettaglio - la definizione dei prezzi minimi garantiti e un regime integrativo dei ricavi degli impianti a bioliquidi sostenibili - che sono tutte misure che devono essere lette nel loro complesso, attraverso una visione che tenga conto della necessità di andare verso la soluzione di un annoso problema che prima di noi

iniziative a favore dell'interesse nazionale. Oggi, finalmente, festeggiamo un sano pragmatismo che cerca soluzioni possibili e praticabili che, pur non promettendo di realizzare il paradiso in terra, garantiscano perlomeno le migliori condizioni di tranquillità verso gli obiettivi della transizione ecologica e anche il rispetto di tutto quel complesso di di impegni a cui l'Italia si è sottoposta a livello internazionale ed europeo, che ci dovranno portare alla decarbonizzazione. Chiaramente non possiamo imporre questo continuando a sacrificare enormi risorse per tamponare la crescita dei prezzi che si riflettono su imprese e cittadini, ma dobbiamo consentire di elaborare strategie che ci portino in tranquillità a finalmente alla sua realizzazione e quindi verso gli obiettivi tanto richiesti e voluti nel contesto europeo. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà. autonomia costituzionalmente garantita, mi limito a osservare come sia ormai evidente il carattere frammentario, confuso e precario della normativa prodotta attraverso gli emendamenti ai decreti-legge e come questa produca difficoltà interpretative e applicative. Tutto ciò acuisce i problemi, allunga i tempi dell'attività dell'amministrazione, disorientando amministratori, cittadini e imprese». Sono le testuali parole con le quali il Presidente della Repubblica ha richiamato una volta di più il Governo e le forze politiche a un dovere di continenza nell'esercizio della decretazione d'urgenza. Parole evidentemente cadute nel vuoto per un Governo che da ultimo, con questo decreto, per l'ennesima volta sottopone al Parlamento un provvedimento mal scritto e mal posto. Siamo di fronte a un testo legislativo confuso, frutto di una sovrapposizione di norme confluite da più decreti-legge, pratica anch'essa più volte stigmatizzata dal Comitato per la legislazione, essendo quello della confluenza cito anche qui testualmente - «un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario *iter* di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari». Siamo di fronte dunque a un'eccezione che è divenuta una regola, che mortifica questa Aula. Devo dire, ancora una volta, che mortifica più la maggioranza delle opposizioni, la quale maggioranza però si fa sempre mortificare volentieri. In definitiva ciò rappresenta, in tutta la sua gravità, quello che il grande senatore e presidente della Corte costituzionale Leopoldo Elia definiva e denunciava come la "fuga dal Parlamento". Questa è la prima fondamentale ragione di critica a questo provvedimento in quanto tale, ma anche come esempio eloquente di un certo modo di governare il Paese e di una modalità inaccettabile di regolare i rapporti di equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo. Purtroppo non è l'unica critica. Infatti, entrando nel merito del decreto, bisogna anzitutto evidenziare che le norme in esso contenute in materia di enti locali e di energia sono insufficienti (e voi lo sapete bene). Sono lacunose e non in grado di assicurare strategicità ed efficacia all'azione di Governo su comparti vitali della vita del Paese a cominciare dalla parte del decreto dedicata alle bollette. Le norme introducono per l'anno in corso nuove risorse per aumentare le soglie ISEE da 20.000 a 30.000 euro, quale presupposto per avere accesso alle agevolazioni riconosciute sulle tariffe delle utenze domestiche. Si proroga inoltre la riduzione IVA al 5 per cento per il gas metano per usi civili e industriali. Queste sono le due misure partorite dal decreto e, quindi, dal Governo. È del tutto evidente che è poco. Davvero non è comprensibile, prima ancora che per ragioni politiche, per mera logica, quali siano le motivazioni per chiudersi al confronto e bocciare tutte le nostre proposte volte a rafforzare la portata sociale del decreto in materia di costi energetici. Vorrei chiedere qui al Governo - per il tramite del Presidente - per quale motivo sono state bocciate le nostre proposte per introdurre crediti di imposta e azzeramento degli oneri di sistema per il settore elettrico, come già previsto in favore del settore del gas. I costi per le bollette elettriche non sono un peso per le imprese al pari di quelli Per quali ragioni, per quali argomenti la maggioranza ha voluto bocciare la nostra proposta di istituire un fondo di 50 milioni per incentivare l'autoconsumo delle piccole e medie imprese, per mezzo di un contributo a fondo perduto per la parziale copertura dell'installazione degli impianti? In base a quale valutazione si è deciso di respingere le nostre proposte a favore degli enti locali, per sostenere le spese derivanti dagli aumenti dei costi energetici, utilizzando ad esempio il fondo crediti di dubbia esigibilità? Come non ho fatto ricorso a un inutile *escamotage* retorico per evidenziare le scelte sbagliate che vi siete arrogati la responsabilità di assumere. Ho fatto vere richieste, che vi pongono di fronte alle vostre scelte o, per meglio dire, alle vostre mancate scelte. Mancate scelte evidenti sul tema bollette e caro energia, come appena detto, ma non meno evidenti sul tema delle infrastrutture energetiche. Anche su questa seconda parte del decreto il Partito Democratico si è assunto l'onere di avanzare proposte concrete, che anch'esse, tra indisponibilità al dialogo e questione di fiducia, sono state respinte da maggioranza e Governo. Avete respinto la proposta del PD di limitare il ricorso a nuovi rigassificatori nei soli casi in cui è a rischio la sicurezza energetica nazionale e questo chiarisce in modo lampante quale sia l'intendimento autentico del Governo: quello di non mettere in campo tutte le azioni possibili per favorire la decarbonizzazione e promuovere convintamente le fonti rinnovabili. Altrettanto eloquente e parimenti non condivisibile è la scelta di respingere la nostra proposta per raddoppiare le misure compensative destinate alle comunità locali, raddoppiando gli indennizzi dall'1 al 2 per cento a valere sul valore complessivo dell'opera. La nostra è una proposta a favore dei territori e della giustizia tra essi, considerato l'onere che alcune Regioni e città si sono assunti in favore dell'intero Paese: ad esempio, l'onere assunto dalla città di Piombino, per il quale abbiamo proposto un fondo da 800 milioni per il rilancio socioeconomico; ma anche questa iniziativa è stata puntualmente bocciata. un'occasione mancata per dare risposta a un pezzo del mondo del lavoro, quello delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle attività connesse al servizio di maggior tutela, recentemente oggetto di decisioni del Governo per il passaggio definitivo al mercato tutelato. Il Governo non sa o finge di non sapere che sono migliaia quelle lavoratrici e quei lavoratori che oggi, con questo provvedimento, avrebbero potuto trovare una risposta alle loro preoccupazioni per il futuro, non solo e non tanto con la proposta del PD - anche questa respinta - di prorogare al 2025 la maggior tutela, dandosi il tempo giusto per immaginare la soluzione, ma attraverso scelte strutturali che a tante professionalità e a un'intera filiera possono garantire una soluzione di lungo periodo, magari attraverso l'applicazione della clausola sociale per la continuità occupazionale, ovvero attraverso altri sistemi di garanzia dei livelli di occupazione e accompagnamento all'interno del mercato del lavoro. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, questo elenco di mancate scelte non è un *cahiers de doléances*, fin troppo facile e scontato, di un parlamentare di opposizione, piuttosto la constatazione evidente che manca una visione prospettica e un progetto per il Paese, in particolare su un tema fondamentale come quello dell'energia. A tale proposito voglio dire che ormai è del tutto evidente - lo dico anche alla mia parte politica - che le destre, soprattutto quelle estreme europee, stanno scegliendo proprio sulle politiche *green* il terreno di scontro privilegiato dei prossimi mesi. L'ha scritto bene di recente Remko Andersen in relazione alla crescita dell'AFD in Germania. Si chiudono non solo gli occhi, ma tutti i sensi, al caldo, ai morti che provoca, alla desertificazione, all'effetto guerra che genera l'effetto serra, alle migrazioni forzate migrazioni forzate di milioni di persone che vengono strumentalizzate quando arrivano in Europa, ma di cui non ci si chiede il motivo per cui scappano dai loro Paesi. "Strumentalizzazione" è la parola centrale, perché si va dalle persone che sono più preoccupate dalla transizione ecologica, in particolare quelle che vivono nelle aree interne, magari gli agricoltori, le persone più fragili, coloro che guardano con preoccupazione alla possibilità che possa aumentare il costo del carburante, che possano perdere un sussidio anche se ambientalmente dannoso. Si va a dire a quelle persone, che sono legittimamente preoccupate, che la transizione ecologica è contro di loro. Così facendo, voi inchiodate il nostro Paese e l'Europa al passato e lo mettete in pericolo, perché sapete come lo tranne i negazionisti - che siamo al centro di un disastro. Certamente noi pensiamo che la transizione ecologica debba essere giusta, solidale, corretta, corretta, che si devono accompagnare con essa le lavoratrici e i lavoratori, ma è anche inesorabile e necessaria: questa è la consapevolezza che noi abbiamo e che voi fate finta di non avere per mere ragioni elettorali, ma di cui - lo voglio dire - vi vergognerete tra qualche anno, di fronte ai disastri che aumenteranno. Investire sulle rinnovabili, sulla decarbonizzazione, su una giusta transizione ecologica, su interventi di *welfare* efficaci contro il caro bollette e su misure per la tutela dei livelli occupazionali connessi al tema energetico: ...*essere contenuto anche in questo testo normativo. Tutto questo invece nemmeno in parte trova accoglimento tra gli articoli e i commi in discussione. Si tratta dell'ennesimo provvedimento con decretazione per necessità e urgenza, ma che di necessario e urgente non contempla le priorità e i bisogni del Paese.

partire da una frase, che penso possa essere comune a tutti, forze di minoranza e maggioranza. Mai più l'Italia dovrà trovarsi in una situazione di fragilità e di esposizione alla variabilità delle dinamiche esterne,

che con questi decreti stiamo ignorando le esigenze degli italiani; voi le avete ignorate per dieci anni e continuate senza rendervi conto di quello che chiedono i cittadini.

come è orgoglioso il nostro Governo di averlo proposto e di portarlo avanti. Signor Presidente, di fronte a uno scenario un un po' tragico direi come quello che ci siamo trovati ad affrontare otto mesi fa - non otto anni fa, ma otto mesi fa - il Governo ha deciso di agire in maniera rapida, improntando però le azioni su una doppia via: ha deciso di muoversi, sia da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista degli investimenti. Se infatti, da un lato, va ad agire con incisività per proteggere e tutelare chi sta subendo le conseguenze economiche più gravi di queste oscillazioni così pericolose, dall'altro lavora affinché l'Italia raggiunga l'obiettivo dell'autosufficienza energetica, quella famosa e tanto decantata dal Governo precedente e mai raggiunta: si parla di percentuali esigue in dieci anni. Proprio qui

potenzialità che purtroppo è stata mortificata da precedenti Governi, ma che ora noi vogliamo assolutamente portare avanti con la massima energia e la massima forza. Gestione delle emergenze, lungimiranza e pianificazione: sono queste le azioni che il decreto

da un punto di vista economico i *bonus* sociali che verranno attuati grazie ad appositi provvedimenti ARERA e i 175 milioni stanziati per eliminare le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri rigenerati dal sistema per i gestori del gas,

tutte grandi azioni per agevolare le famiglie che oggi risentono di più di questa grave crisi energetica. Voglio però soffermarmi sul grande tema della lungimiranza, perché finalmente abbiamo un Governo che vede oltre

piacere solamente al cittadino per ottenere i voti alle prossime elezioni comunali, regionali o politiche. Governo ha fatto sul tema dei rigassificatori, di cui tanto si sta parlando, è unico, è veramente una cosa da segnare: peccato che i giornali abbiano poco esaltato il grande lavoro fatto dal Governo.

Il Governo qui ha affrontato, con coraggio, le preoccupazioni che arrivavano dal territorio e dai sindaci, ascoltandoli per interi mesi. Hanno lavorato insieme e hanno trovato soluzioni, non solo da un punto di vista economico ed energetico, ma anche di amore e di rispetto per il territorio e la qualità vita dei cittadini che lo abitano. Piombino è l'esempio eclatante: la città è stata protagonista di attività di rigassificazione delle quali poi beneficeranno tutti gli italiani.

voi, che ci fate una lezione quotidiana sull'ambiente. Questo decreto introduce la VIA, la valutazione di impatto ambientale, portando i famosi centoventi giorni per il rilascio dell'autorizzazione a guardate che non si aumenta il tempo, ma lo si diminuisce, perché in questo modo evitiamo ricorsi, comitati del no e una serie di problematiche, perché la VIA permette finalmente di capire se quel posto è idoneo o no.

di cui ho parlato fino ad ora era ben noto all'amministrazione regionale, che è, sì, di sinistra, ma si vede che in quel momento non interessava ascoltare un sindaco che era dell'altra parte politica.

il punto è che noi siamo per i fatti. Siamo per la vera tutela ambientale, in risposta ai vuoti *slogan* dell'opposizione. Siamo per un'Italia finalmente cuore pulsante del Mediterraneo e *hub* energetico indipendente, forte e libero dai condizionamenti esterni e dalle direzioni ambigue delle varie dinamiche internazionali. Non voglio chiudere con uno *slogan* dei nativi americani, americani, che poi ho visto in una grande catena di pizzerie. Voglio chiudere con lo *slogan* degli italiani, quelli che tutti i giorni ci chiedono, quando ci incontrano fuori: aiutateci. Governo, aiutaci. E noi di Fratelli d'Italia, insieme a tutti i colleghi della maggioranza, siamo fieri di ribadire, anche in questa occasione, la nostra piena fiducia al Governo e a questo decreto. Soprattutto, vogliamo dire agli italiani che ci siamo. E gli italiani ci stanno ripagando, come dicono i sondaggi. *(Applausi)*.

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che approviamo oggi definitivamente è stato necessario ed urgente per intervenire sostanzialmente su tre filoni: le disposizioni per le Regioni a statuto ordinario in materia di sanità, le disposizioni per garantire la tempestiva attuazione del PNRR, in particolare per assicurare la parità dei sessi nelle gare pubbliche e per favorire l'edilizia universitaria

Le norme al riguardo mirano a difendere l'interesse nazionale dell'Italia e a raggiungere l'indipendenza energetica del Paese, attraverso il il proseguimento e l'implementazione della politica sulla diversificazione dell'approvvigionamento delle diverse fonti energetiche. È una politica che sta già dando i suoi frutti, consentendo all'Italia di non dipendere più dal gas russo, cosa che avverrà in maniera totale e definitiva entro pochi mesi. In tal senso, il rigassificatore già in funzione a Piombino sta dando il suo importante contributo. Si tratta di una scelta lungimirante, che non posso non sottolineare ancora una volta con grande favore. Nel decreto-legge, come accennavo, sono contenute misure di semplificazione importanti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione sia per la loro futura ricollocazione, insieme a norme tese a garantire procedure chiare e veloci per l'entrata in funzione di una nuova capacità di rigassificazione, consentendo di evitare future criticità energetiche. insomma, di un provvedimento tutto volto alle necessità concrete dell'Italia di fronteggiare la crisi energetica, dovuta essenzialmente al conflitto in atto da più di un anno in Ucraina.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, oggi l'Assemblea si impegna a ratificare l'ennesimo provvedimento *patchwork* su un settore strategico per il Paese, quello energetico, le cui difficoltà, negli ultimi anni, hanno messo a dura prova la capacità di resistenza economica di cittadini e imprese. un tema cruciale, su cui ancora una volta l'Esecutivo ha deciso di porre irresponsabilmente il voto di fiducia, impedendo che si realizzassero le condizioni minime per instaurare un serio e necessario dibattito parlamentare. Lo vorrei ricordare alla presidente Meloni, la quale si era pubblicamente impegnata, nel gennaio scorso, a ridurre il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza, strumento che - anche a detta sua - esautora e mortifica la capacità deliberativa del Parlamento. avvilente rendersi conto che la parola data valga quanto un due di picche. Nello specifico, il disegno di legge in esame introduce la possibilità di realizzare nuova capacità di rigassificazione fossile, senza tuttavia tenere minimamente conto del reale impatto economico, sociale e ambientale degli interventi incentivati. È questo il classico approccio metodico a cui il Governo in carica ci ha purtroppo abituati e che rispecchia la dichiarata visione politica dell'Esecutivo, che ritiene il combustibile fossile gas una priorità per la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica. Così, ancora una volta, ci troviamo qui a chiederci come sia possibile non considerare le ricadute prodotte dai rigassificatori sulle dinamiche del mercato elettrico, sulla fattibilità economica e sui gravi e non più sostenibili danni ambientali derivanti dall'utilizzo delle fonti energetiche fossili e dei loro effettivi impatti. Possibile che, a fronte di tutti gli eventi climatici estremi che stanno mettendo in serio pericolo la qualità di vita di cittadini, creando ingenti danni alla nostra economia, si debba ancora stare a discutere se la crisi climatica esista o no o se abbia senso la transizione ecologica? Possibile che non si passi alla fase successiva, quella di rimboccarsi le maniche e affrontare seriamente la messa in sicurezza dell'Italia, con solidi provvedimenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione del dissesto idrogeologico? Il nostro Paese, sottoscrivendo il raggiungimento degli obiettivi climatici, sia a livello internazionale sia europeo, ha accettato questa importante sfida. Il Governo Meloni invece, sordo a tutti gli appelli della comunità scientifica e ai reali interessi di questo Paese, sta facendo di tutto per rallentare questa corsa. Ricordo che il pacchetto europeo Fit for 55 e la comunicazione REPower EU chiedono agli Stati membri uno sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per cento del *mix* energetico a livello europeo al 2030; un incremento dell'efficienza energetica sul consumo finale di energia al 2030 e una ristrutturazione in chiave di efficienza di circa il 25-30 per cento degli edifici al 2033. Lo chiedono per abbattere le emissioni climalteranti, non per il semplice gusto di vessare i propri cittadini. Queste misure servono per garantire un presente e un futuro migliore all'Italia, al nostro pianeta e alle persone che lo abitano. Intanto, placidamente, il Governo bypassa tutti gli impegni presi, concentrato com'è nel rendere l'Italia e il Mediterraneo un *hub* del gas, un'azione antieconomica e controproducente tanto per gli impatti ambientali, quanto per quelli sanitari e sociali. Non rientra infatti nelle sue corde - l'ha detto più volte - trasformare l'Italia in un *hub* verde, puntando su energia rinnovabile, su sole ed eolico, su reti elettriche, accumuli ed efficienza energetica, materiali e prodotti per l'uso circolare, circolare, oltre alla messa in sicurezza degli ecosistemi naturali e della biodiversità. Questo sì che garantirebbe la costruzione di un futuro ambizioso e sostenibile, anche economicamente e in termini di vero risparmio sulle bollette. Perseguendo una precisa logica politica, questo disegno di legge, da un lato, prevede opere per l'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, dall'altro, getta fumo negli occhi ai cittadini, offrendo loro un irrisorio segnale di apertura al sostegno dell'autoconsumo energetico. Così facendo, tale provvedimento tenta malamente di rendere credibile un dispositivo che non si allinea in maniera adeguata al raggiungimento del taglio delle emissioni di gas effetto serra, responsabili dell'aumento della temperatura che causa gli eventi climatici estremi, e all'obiettivo di neutralità climatica. Puntare ancora su nuovi impianti alimentati a gas fossile non permette la concreta realizzazione di un piano per l'efficienza energetica e non agevola lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile nel settore industriale. industriale. Sarebbe auspicabile utilizzare bene e meglio i fondi e le risorse economiche del PNRR per traguardare lo scenario di decarbonizzazione previsto nella bozza del Piano nazionale integrato energia e clima. Gli obiettivi climatici europei al 2030 implicano per l'Italia una produzione elettrica rinnovabile di circa il 70 per cento rispetto all'attuale 35-40 per cento, per raggiungere un sistema elettrico prevalentemente decarbonizzato nel 2035, come da impegni del G7. Ribadiamo con forza che l'Italia non ha bisogno di nuove infrastrutture, gasdotti e rigassificatori per coprire il fabbisogno energetico nazionale e che può dimezzare e progressivamente eliminare la dipendenza dal gas fossile attraverso un *mix* di energie da fonti rinnovabili, risparmio energetico, efficienza energetica e sfruttamento delle infrastrutture esistenti, obiettivi che possono essere parzialmente traguardati anche per mezzo di azioni immediate di risparmio sui consumi che andranno a beneficio delle tasche degli utenti. Ai risparmi ottenuti nel breve periodo si aggiungerebbero anche i notevoli risparmi ottenuti, per esempio, da maggiori investimenti strutturali sulle comunità energetiche rinnovabili e sulla rete elettrica.

Per contro, bisogna smettere di perseguire costose politiche energetiche che, con gli attuali prezzi di mercato, i consumatori non possono più sostenere economicamente. Riguardo alle politiche su clima e transizione energetica va perseguita l'installazione di nuova capacità da fonti di energia rinnovabili, passando anche da tecnologie alimentate a gas a quelle alimentate a elettricità, ad esempio da caldaia a gas a *boiler* elettrico. Ciò ridurrà sostanzialmente il consumo di gas in Italia e in Europa, facendo risparmiare ulteriormente i cittadini italiani. Insistere sulla rigassificazione, come il provvedimento in discussione si propone di fare, comporta inoltre il rischio di vincolarci in modo non auspicabile a livello geopolitico. Nell'ambito del mercato unico e interconnesso europeo è impensabile immaginare un uso autarchico dell'energia: anche nella prospettiva di diventare un *hub* di transito del gas verso l'Europa centrale, costruire infrastrutture dai costi elevati in Italia significa pagare un alto un alto prezzo per una capacità di importazione per il mercato europeo che non avrebbe senso economico, dal momento che anch'esso è in fase di veloce trasformazione. Il costo di nuove infrastrutture e forniture alimentate a gas fossile, oltre agli elevati impatti dannosi per l'ambiente e la biodiversità, sarebbe finanziato principalmente dalle bollette delle famiglie e delle imprese. Più appropriata, invece, risulterebbe l'intenzione di destinare maggiori risorse economiche agli interventi di efficienza energetica, così da rendere chiara la convenienza economica dell'utilizzo delle energie rinnovabili rispetto a quelle fossili. Quel che di certo si può dire è che saranno i soli contribuenti a pagare per intero sia i costi delle nuove infrastrutture sia gli impegni commerciali di approvvigionamento di lungo periodo sottoscritti in qualunque forma dallo Stato. Infatti, dal momento che il gas viene acquistato dalle aziende e non dai Governi, ogni qualvolta un Governo fornisce garanzie ad accordi commerciali si espone a rischi di aiuti di Stato e in generale a conflitti di interesse e opacità nei meccanismi decisionali. Tale rischio si accentua quando il Governo è azionista delle aziende interessate. In termini di rischio climatico, qualunque impegno sui combustibili fossili che sia un contratto di lungo periodo su un'infrastruttura prolunga dannosamente la nostra dipendenza dal gas fossile. Tale scelta rallenterebbe le politiche di decarbonizzazione, portando ad un contemporaneo aumento dei prezzi energetici e delle emissioni climateranti. Tutto questo sulle spalle dei cittadini.

Signor Presidente, il decreto-legge in esame ha mutato la propria composizione iniziale: i primi due articoli, che riguardavano gli enti territoriali, sono già confluiti in un altro provvedimento il nuovo testo, già approvato dalla Camera, è diventato uno strumento strategico per la produzione di energia in Italia. Lo è, a maggior ragione, data la necessità di cambiare la tipologia e la natura degli approvvigionamenti energetici dopo la rottura delle relazioni con la Russia conseguente al conflitto in Ucraina. Ovviamente non eravamo i soli in Europa a dipendere dalle forniture della Russia, posto che ad esempio la Germania sta subendo più gravi conseguenze. Era talmente conveniente produrre energia dal gas russo, talmente a buon mercato, che persino l'energia prodotta dagli impianti solari del nostro Paese entrava in rete dopo aver utilizzato il gas. Ora si è dovuto attuare un totale cambio di paradigma, mettendo al primo posto l'energia da noi prodotta e agevolando ovunque possibile la produzione nazionale. Nel frattempo, verrà utilizzato anche il gas proveniente da altri fornitori, che, avendo un costo maggiore, cui si aggiunge quello della rigassificazione, dovrà poi essere gradualmente integrato Nel provvedimento sono presenti norme puntuali per consentire ai rigassificatori come quello di Ravenna di essere pienamente operativi. Riteniamo che la strategia messa in atto dal ministro di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin per conto del Governo Meloni rappresenti un punto di svolta strategico verso la sicurezza energetica, avendo ben chiaro l'obiettivo finale dell'indipendenza energetica, una strategia che ci consentirà in tempi brevi un marcato ridimensionamento della dipendenza dalle forniture estere. L'idea di puntare in modo deciso sulle energie alternative e sulle rinnovabili rappresenta il punto di svolta anche nelle modifiche introdotte alla Camera: dall'utilizzo del fotovoltaico alla valorizzazione delle biomasse all'uso del geotermico all'impiego del biometano. L'introduzione di ulteriori procedure semplificate agevolerà la costruzione e l'utilizzo di nuovi impianti. Sono previste procedure abilitative semplificate per la riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Inoltre, anche gli interventi per la produzione di biometano già in funzione possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata. Sono previste disposizioni per efficientare le infrastrutture strategiche del nostro Paese, cioè appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e degli oleodotti delle principali direttrici o corridoi infrastrutturali, per le quali sono previste procedure autorizzative più veloci. Il decreto contiene inoltre il rinnovo dei cosiddetti *bonus* sociali, cioè il riconoscimento delle agevolazioni per la luce e il gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, così com'è stato confermato l'azzeramento, sempre per il terzo trimestre di quest'anno, delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Inoltre, vi è la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali, allargando questa volta la stessa aliquota anche al teleriscaldamento. di un pacchetto di *bonus* che hanno l'obiettivo di continuare a sostenere famiglie e imprese, così com'è stato fatto dall'inizio del Governo Meloni, misure che hanno evitato il fallimento di migliaia di imprese e hanno aiutato decine di migliaia di famiglie a continuare a fruire di servizi essenziali quali il riscaldamento e la luce elettrica. Il decreto mette insieme una serie strutturata di misure che seguono quel filo logico di dare una più puntuale valorizzazione alle nostre energie e alle fonti necessarie per produrle. Con questa legge, l'indipendenza e la sicurezza energetica sono più vicine, un altro passo di un cammino che vogliamo percorrere fino in fondo. C'è chi arringa parlando di decreto farsa, di decreto vuoto, c'è chi promette grandi e utopiche rivoluzioni *green* e poi ci siamo noi, che lavoriamo per realizzare i nostri programmi e aiutiamo il Paese a uscire dalla crisi energetica. Forza Italia e il centrodestra con questo provvedimento dimostrano gli italiani di saper trasformare le parole in fatti e per queste ragioni annuncio il voto favorevole alla fiducia dei senatori di Forza Italia.

da non sentire il bisogno di confrontarvi con il Parlamento. Eppure, siamo in una democrazia e, per quanto a voi la cosa possa sembrare una noiosa e tediante perdita di tempo, i provvedimenti devono seguire un *iter* obbligato, pensato proprio per evitare che in pochi possano prendere decisioni basate esclusivamente sul sentire di una sola parte politica. "Ma noi abbiamo vinto le elezioni" è la vostra ostentazione più gettonata. Certo, Certo, le avete vinte, ma mi permetto di ricordarvi che le avete vinte in un sistema che al momento è ancora parlamentare e che, per di più, ha al suo centro proprio i due rami del Parlamento, che, con il vostro atteggiamento, sembrate voler recidere o quantomeno mortificare nelle proprie funzioni e prerogative. Alla luce del testo che ci proponete, sento di chiedervi se avete letto il provvedimento prima di approvarlo in Consiglio dei ministri. Il mio è un dubbio legittimo. Non me ne voglia il ministro Sangiuliano, ma spero che in Consiglio dei ministri non sia valsa la prassi del premio Strega, secondo cui si può votare un testo senza sapere di cosa parla. Ennesimo decreto, quindi, che arriva all'esame di quest'Assemblea dopo giorni segnati da dichiarazioni di alto livello intellettuale, politico e morale, spesso rilasciate ad arte da esponenti della maggioranza e gregari simpatizzanti, forse con il solo intento di distrarre, tuttavia frutto di sincero sentire, e in ogni caso imbarazzanti. Questo Esecutivo si mostra privo di strategia energetica e climatica e, allo stesso tempo, molto attento agli interessi degli operatori del fossile. Nel testo semplificate ulteriormente sia le procedure autorizzative ambientali per la realizzazione di nuovi e inutili rigassificatori galleggianti, sia gli *iter* autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture considerate strategiche appartenenti alla rete dei gasdotti e degli oleodotti. Insomma, anche questa volta avete adottato una serie di scelte costose, che garantiscono risorse ai privati per il ritorno dei loro investimenti, scaricando tutti i costi sulla collettività, attraverso il pagamento delle prossime bollette. In questo modo, senza alcun rischio di impresa, è facile farla l'impresa, socializzando i costi e privatizzando gli utili. Tutto questo avviene in uno specifico scenario, in cui gli approvvigionamenti dalla Russia sono ormai pochissimi e gli stoccaggi sono quasi pieni. Teniamo presente che in Italia sono stati risparmiati circa 10 miliardi di metri cubi di gas in otto mesi, pari a una riduzione del 18 per cento dei consumi. Nel 2022 abbiamo consumato 68 miliardi e mezzo di metri cubi di gas, ovvero 7 in in meno rispetto al 2021. La disponibilità di gas però è rimasta la stessa: 75 miliardi di metri cubi, pari a quella del 2021, mentre ad aumentare del 200 per cento sono stati solo i metri cubi di gas esportati. Per il resto, questi numeri ci dicono che l'attuale sistema delle infrastrutture energetiche garantisce il dovuto approvvigionamento. Allo stato attuale, i rigassificatori di Ravenna e Piombino (quest'ultimo, tra l'altro, collocato in un'area di crisi complessa) sono ininfluenti ai fini della sicurezza energetica e servono soltanto a consolidare la narrazione del Governo e quindi del presidente Meloni, ma anche della stessa Snam, nel fare dell'Italia l'*hub* del gas del Mediterraneo. Nel frattempo, i colossi dell'energia collezionano extraprofitti da capogiro, che non vengono tassati, e la transizione energetica verso le rinnovabili resta ferma resta ferma al palo ovvero si muove a passo di lumaca. *(Applausi)*. Anche le associazioni del settore ci dicono che in soli tre anni con eolico e fotovoltaico si possono ottenere 60 gigawatt, ma, ogni volta che si tenta un approccio ecologico al tema dell'energia, dal Governo Meloni si grida all'ambientalismo ideologico. Così, mentre tutto il mondo aumenta i propri sforzi per arginare i cambiamenti climatici e le tossicità l'Italia resta ferma e imbalsamata. Colleghi, i rigassificatori sono ininfluenti per la sicurezza energetica del Paese e il decreto in questione è l'ennesima prova della volontà del Governo di svuotare il ruolo del Parlamento, visto che ci si è di nuovo affidati a una decretazione d'urgenza che nulla ha a che vedere con la materia in esame. Il Governo dovrà assumersi tutta la responsabilità di questa scelta. In questo quadro, molto probabilmente aumenteranno i costi per l'energia, già attualmente elevati, senza beneficio alcuno e mettendo a rischio anche la competitività delle imprese del nostro Paese. Anche con questo provvedimento quindi continuate ripetutamente a strizzare l'occhio alle fossili, mentre a tutte le proposte che abbiamo avanzato in Commissione avete risposto risposto di no *a priori*, senza alcuno scambio di vedute o punti di vista. Che le opinioni altrui siano invise a questa maggioranza è un dato di fatto che non scopriamo di certo oggi, ma mi chiedo dove vi porterà questo atteggiamento. Questo provvedimento arriva alla fine di una settimana strepitosa, fatta di fantastiche esternazioni e prese di posizione da parte di diversi esponenti del Governo. credo sia il trentesimo decreto-legge: per molto meno, in una situazione ben diversa, avete definito criminale il presidente Conte *(Applausi)*, occupato a contrastare una pandemia. A proposito, stranamente pare che nessuno di voi sia più andato a fare benzina, dopo il fortunato *spot* elettorale: non vi siete accorti dei nuovi aumenti? Certo, evidentemente i vostri problemi oggi sono altri. Il fatto è che siete a secco di idee e programmi, e questa è la verità. Per mascherare la vostra manifesta inadeguatezza, provate a distrarci con esternazioni deliranti che, nel vostro caso, non possiamo neanche attribuire al caldo di questi giorni, visto che per molti di voi i cambiamenti climatici non esistono. *(Applausi)*. Signori del Governo, dove sono i 1.000 euro promessi ad ogni cittadino con un semplice *click*? Cosa ne è stato del blocco navale a suo tempo tanto facile da attuare? Dov'è la riduzione delle accise? accise? Siete il Governo del sì e no, a testimonianza del fatto che non siete quasi mai convinti di nulla e che state procedendo per tentativi e senza alcuna alcuna visione. Abolite il superbonus, ma riscrivete il PNRR per rifinanziarlo; abolite il reddito di cittadinanza, ma non del tutto; date alle persone in difficoltà un euro al giorno per comprare il pesce fresco, ma siccome siete sotto pressione vi dimenticate di inserire il sale nella lista. Il Ministro della giustizia dice di voler cambiare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, perché per lui è evanescente e non esiste, ma poi vi ricordate di avere Paolo Borsellino nel vostro *pantheon* e cambiate idea. Su una cosa - e di questo bisogna darvi atto - invece siete abbastanza decisi e continuate a strizzare l'occhio agli evasori, passando dal pizzo alla prigione di Stato. Siccome ci tenete tanto a fare le cose perbene, alla Camera bocciate la direttiva europea sulla lotta alla corruzione,

parlano da soli e ci raccontano di un Esecutivo ancora in cerca d'autore. È il Paese che dicevate di voler prendere per mano, non Joe Biden. Siete totalmente inadeguati quanto pericolosi, e questa cosa ce la ricordate voi stessi giornalmente. Signor Presidente, per questo, ma anche per tanti altri motivi che non sto qui a dire, dichiaro il voto contrario a questo provvedimento da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

come legislatori, oggi siamo chiamati a occuparci di materie vitali per il Paese e per le famiglie, in un momento particolarmente complicato della nostra storia e della nostra quotidianità.

Eppure il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire, come sappiamo, è incentrato su provvedimenti in tema di energia che hanno due obiettivi primari: uno di respiro immediato, continuare ad aiutare le famiglie e le imprese in questa fase difficile sui costi energetici, e l'altro di respiro molto più ampio, anche se più lungo, portare l'Italia a raggiungere finalmente l'indipendenza in campo energetico. Già solo l'enunciazione di questi princìpi che stanno alla base del decreto-legge e ispirano la nostra azione di Governo dovrebbe spingere le opposizioni a sposare in tutto o in parte le nostre scelte, che sono indiscutibilmente e indubbiamente compiute nel solo interesse del Paese e dei nostri concittadini. Invece, questo non è. I colleghi ci criticano, dimostrando di aver evidentemente già dimenticato quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, i cui strascichi ancora ci portiamo dietro, e quante quante preoccupazioni ci hanno angosciato; hanno già dimenticato come la situazione geopolitica internazionale abbia fatto emergere con tutta la sua dirompenza proprio la nostra vulnerabilità,

come questa dipendenza e questa vulnerabilità dell'Italia siano dipese proprio da alcuni di loro. Mi riferisco innanzitutto ai colleghi del PD, responsabili per primi di averci consegnati mani e piedi alla Russia e ad altri Stati per la fornitura di gas ed energia e di averci posto in una situazione di subalternità quale nulla hanno poi fatto per tentare di farci uscire, se non adesso, rigirando le carte in tavola per far apparire noi come quelli che vogliono ricarbonizzare la Nazione a danno di tutti. Questo non è il modo migliore per celare le vostre malefatte. Non siete voi forse quelli che, mascherandosi dietro un ecologismo di facciata, hanno votato in Europa per l'abolizione dei veicoli a combustione, con un miope integralismo elettrico che non fa che consegnarci dalla Russia alla Cina, per di più con un danno di sproporzioni smisurate per la nostra economia e, soprattutto, per le fasce meno abbienti della nostra popolazione? Ribadisco che, se siamo in questa situazione così critica anche in materia energetica, la responsabilità non è certo la nostra. Anche stavolta siamo chiamati a porre rimedio ai danni che voi avete fatto a causa della vostra incapacità, delle vostre scelte scellerate e, soprattutto, del vostro In ogni caso, le cose di cui ci accusate sono menzogne, perché con questo decreto introduciamo innovazioni molto coraggiose, con le quali buttiamo le fondamenta

di cui dobbiamo servirci da qui ai prossimi anni. Dovremo certamente pian piano abbandonarli, ma solo attraverso un piano energetico che guardi certamente al sole, al vento, all'acqua e alla geotermia, ma soprattutto al nucleare di nuova generazione e da qualche parte bisogna pure iniziare e partire. noi ci assumiamo l'onere di farlo, nel modo, credo, più razionale possibile, scegliendo ciò che può avviare questo percorso in tempi rapidi, con una semplificazione normativa che il Governo e la Lega in particolare perseguono fin dal primo momento, offrendo assoluti benefici per i cittadini, che finalmente possono creare sviluppo, ottenere risposte alle loro istanze e realizzare anche le proprie ambizioni, senza venire risucchiati da cavilli e da blocchi degli *iter* amministrativi che portano solo a fermare la crescita. tuttavia, che chi come voi è stato il primo colpevole dell'estrema burocratizzazione dello Stato di quest'opera di semplificazione non possa certo oggi gioire, perché significa perdere potere, il potere che nasce dalla creazione del bisogno. Noi, invece, andiamo avanti proprio su questa strada, perché è l'interesse pubblico che ci sta sempre a cuore. In tema di energia partiamo dalla previsione di più tempo e più possibilità per autorizzare nuovi rigassificatori, con procedure più rapide e più semplici, ma anche più complete, con l'integrazione della via che finora non era prevista e che è il segno tangibile dell'attenzione che abbiamo e riserviamo verso l'ambiente, ottenendo peraltro immediata risposta da parte di numerosi enti territoriali, a dimostrazione, da un lato, di quanto una previsione del genere fosse attesa dai territori come preziosa fonte di approvvigionamento, di risoluzione dei problemi e di ricchezza e, dall'altro, di quanto siamo stati capaci anche in questa occasione di raccogliere interpretare le esigenze dell'Italia. E, soprattutto, andiamo a occuparci di biomasse, incentivandole attraverso l'innovazione di carattere fiscale; di geotermia, con la possibilità di presentare istanze per potenziare gli impianti; e di biometano, con procedure abilitative semplificate e la possibilità di ampliare del 50 per cento la base dell'area dedicata alla digestione anaerobica. tutti provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con il carbone e che dunque smentiscono le vostre menzogne e accuse, andando piuttosto ad aprire finalmente la strada strada a un'indipendenza energetica del nostro Paese, obiettivo cui crediamo possa contribuire, per esempio, anche la possibilità di assimilare agli enti del terzo settore le imprese che si riuniscono in forma di comunità energetiche. È questa una previsione fondata sul mutualismo la cui bontà, dunque, dovrebbe essere essere apprezzata e riconosciuta proprio da chi del mutualismo e della cooperazione ha fatto una bandiera, anche se, in realtà, questo mutualismo lo ha poi usato in modo distorto, come strumento di potere e per lucrare, a volte anche in maniera illecita. A tutto A tutto questo, poi, affianchiamo le politiche di sostegno a chi ha ancora più bisogno. Non dimentichiamo infatti le famiglie svantaggiate, che continuiamo ad aiutare, estendendo le previsioni precedenti e, anzi, rafforzandole con un corposo intervento anche sociale, cui dà vita proprio quella destra che voi, falsamente e continuamente, tacciate di disumanità e disattenzione per i deboli. Concludo rispondendo a un'ultima e ulteriore critica, quella di aver fatto ricorso alla fiducia. Non sto qui a ricordarvi

dell'utilizzo della fiducia dei Governi a trazione sinistra. Non ci fate ridere con le vostre contestazioni, che nascondono il vuoto delle vostre osservazioni. Non avete appigli seri e di contenuto per attaccarci sul provvedimento oggi in approvazione

si occupa di diversi argomenti e in particolare di bollette e rigassificatori; quindi, di costi e fonti dell'energia. Si tratta di questioni molto serie e prioritarie, accorpate per causa del vizio inguaribile dell'Esecutivo Meloni, che arriva in ritardo su tutto e corre soltanto se deve colpire e recidere lo stato sociale, la libertà di dissenso e le tasche degli italiani. È l'ennesimo provvedimento di un Governo ambiguo, che ieri predicava bene e oggi razzola male; che a parole si dice vicino alle famiglie, ma poi non affronta i problemi urgenti e persegue, ostinatamente, a spaccare il Paese e nella destrutturazione dell'unità nazionale, con la responsabilità di forti ritardi circa gli obiettivi di cui al pacchetto energia e clima 2030 e al relativo Piano nazionale. Non parliamo poi dei ritardi complessivi legati al PNRR, dove si sta chiarendo, proprio in questi giorni, l'inadeguatezza del Governo, con il grido di dolore del terzo settore che chiede di essere ascoltato sulla rimodulazione del PNRR; l'abbandono e l'isolamento degli amministratori locali, la totale non chiarezza del ministro Fitto rispetto alle scadenze e alla rimodulazione dei progetti. Questa dovrà avvenire entro il 31 agosto e ancora chiediamo che il Parlamento venga a sapere come il Governo vuole rimodulare e in che modo l'Italia vuole competere sul PNRR: niente di tutto questo. Alla Camera il Governo aveva posto la questione di fiducia su questo decreto, a riprova, semmai ce ne fosse bisogno, della paura della legislazione democratica, che turba e inquieta l'Esecutivo Meloni e la sua maggioranza, che si allinea sempre d'ufficio. Per inciso, con più di trenta decreti in meno di nove mesi, il Governo Meloni ha l'infelice primato della decretazione d'urgenza a colpi di fiducia. Questo modo di agire mortifica il Parlamento e la qualità delle leggi dello Stato, data la grave mancanza del confronto in ambito legislativo, che è quello della rappresentanza, del dibattito, dello scontro politico, ma che è anche quello della sintesi per il bene del Paese. Vorrei appena ricordare che, quando stava all'opposizione, l'onorevole Meloni auspicava un'ampia dialettica sulla conversione dei provvedimenti del Governo. Oggi invece ha dimenticato in fretta quelle sue posizioni, facendo agli altri ciò che non voleva fosse fatto a lei. Ma questa è una caratteristica del presidente Meloni, dei Ministri in carica e dell'intero centrodestra, che proprio sulle bollette dava lezioni morali e oggi tace, come imbavagliato. D'altronde, state di fatto istituzionalizzando un monocameralismo silenzioso, che svilisce il ruolo del Parlamento. Nello specifico, il provvedimento in questione prevede inadeguate e temporanee misure di sostegno per famiglie e imprese rispetto ai costi dell'energia. Infatti, sulle tariffe di corrente e gas, il provvedimento contempla che le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute siano rideterminate dall'ARERA, ma nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023. Nella misura sono inclusi gli effetti derivati dall'estensione della soglia ISEE, da 20.000 a 30.000 euro, volti a consentire l'accesso da parte dei nuclei familiari numerosi al *bonus* sociale legato al disagio economico. Tutto questo significa che i benefici saranno ridotti e brevi, per dirlo in termini spiccioli e comprensibili. Ciò vuol dire che non c'è stata la volontà di un intervento strutturale del Governo, già passato alla storia come l'Esecutivo dell'incoerenza e della propaganda politica. Anche per un elemento di chiarezza da parte nostra, quanto alle misure sui rigassificatori, che il Partito Democratico ha voluto, in una logica di unità nazionale, di diversificazione delle fonti energetiche e di decarbonizzazione, sia per limitare la spirale dei prezzi e per supportare l'Ucraina, sia per indirizzare il Paese verso la transizione verde, il provvedimento è monco per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che concorrono all'obiettivo dell'autosufficienza energetica, che sposammo responsabilmente nel Governo Draghi. Tra l'altro, avevamo proposto di aumentare il sostegno a Piombino e a Ravenna, che ospiteranno queste strutture, ma non siamo stati ascoltati. Inoltre, in questo decreto-legge si potevano azzerare i costi di gestione, anche per la spesa energetica e non soltanto per quella del gas. Ancora, si potevano prolungare i crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, a favore delle imprese energivore o meno. Abbiamo chiesto di raddoppiare le misure compensative destinate alle comunità locali, ma avete detto no. Da questo punto di vista, il Governo si è chiuso e non ha voluto ascoltarci. Il Partito Democratico, con grande senso di responsabilità, ha presentato le sue proposte per migliorare questo provvedimento, ma avete continuato a dire no. In Italia si usa il gas per produrre il 60 per cento dell'energia elettrica. Ciò significa che questo provvedimento, così come concepito, rischia di portare un rincaro strutturale delle bollette, in quanto non contempla le misure sulle rinnovabili, che sarebbero state possibili e più che opportune. il provvedimento di cui stiamo parlando è caotico, scritto male, privo di soluzioni strutturali al caro energia e completamente omissivo sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, esso rischia di portare un aggravio ulteriore e forte dei costi per le famiglie e non darà dei benefici ai cittadini con difficoltà economiche o con problemi di salute.

questione di fiducia sul provvedimento in esame. Voteremo dunque contro, anche nel merito, perché è un provvedimento che ci riporta indietro di anni, ci allontana dal futuro dell'Unione europea e dall'obiettivo della transizione ecologica transizione ecologica *(Applausi)*, su cui si fondano la ripresa e la resilienza collettiva, soprattutto quella delle nuove generazioni. Ci tengo a sottolineare, concludendo, per quanto ci riguarda, noi continueremo a batterci in tutte le sedi politiche per il sostegno alle famiglie, per la diversificazione delle fonti energetiche, per la transizione ecologica e per il rispetto, Presidente, della democrazia parlamentare che il Governo sta calpestando, non considerando i bisogni della persona umana, i diritti dei cittadini, le esigenze della comunità nazionale e il cammino corrente che tutti noi dobbiamo fare per l'unità vera dell'Europa. Per tutto questo dichiaro che il Gruppo Partito Democratico voterà no alla fiducia al Governo. con questo provvedimento si aggiunge un nuovo importante tassello al grande lavoro svolto in questi mesi dal Governo e dalla maggioranza sul tema dell'energia e su quello del sostegno alle imprese e ai cittadini rispetto al tema dei costi delle bollette, anche nell'ottica degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolar modo, attraverso l'esame della Camera dei deputati, sono state introdotte a questo provvedimento norme relative al contenimento dei prezzi nel settore elettrico e di quello del gas naturale. Tra i molti interventi voglio ricordare quelli sul tema della capacità di rigassificazione nazionale, nazionale, fondamentale nella strategia di diversificazione delle fonti e di sicurezza energetica nazionale. In questo senso, viene ampliata la possibilità per gli operatori di presentare nuove istanze ai commissari straordinari e, soprattutto, si prevede che venga razionalizzata la fase autorizzativa, con un procedimento unico che semplifica e allo stesso tempo rende più rigorose le valutazioni ambientali. Questo metodo corrisponde peraltro proprio alla nostra visione sul tema dei procedimenti autorizzativi: se vuoi realizzare un impianto, il decisore pubblico ti deve dire, in tempi certi, se quell'impianto può essere realizzato, se quell'impianto ha bisogno di modifiche, ma di sicuro non ti può rendere ostaggio della burocrazia. Viene poi esteso ai commissari, che ricordiamo sono i Presidenti delle Regioni Toscana ad Emilia-Romagna - a questo proposito la collega Petrucci ha ampiamente ricordato la questione di Piombino e le sue caratteristiche storiche - anche le sue caratteristiche storiche - anche il tema dell'incremento della capacità di rigassificazione; quindi non solo dell'installazione, ma anche delle fasi successive. Sono previsti obblighi sacrosanti di trasparenza e di informazione per le comunità locali, che devono essere coinvolte in questi processi e informate; devono conoscere le questioni e avere le adeguate garanzie, nonché le adeguate compensazioni. Importante in questo senso è anche l'obbligo per i concessionari di manutenzione delle infrastrutture, anche in caso di ricollocazione delle unità galleggianti. Il piano di rigassificazione viene poi inserito nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, proprio perché è necessario avere una visione d'insieme dal punto di vista della strategia energetica. Vi è poi la parte relativa alle bollette, che è un ulteriore intervento per agevolazioni ai soggetti svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e per quelli in gravi condizioni di salute. Da questo punto di vista, mettiamo Da questo punto di vista, mettiamo in campo 285 milioni: questo è un ulteriore intervento, perché ricordiamo che fin dal suo insediamento il Governo è intervenuto nettamente a sostegno delle categorie che avevano necessità. Anche oggi che c'è una fase di crescita, sicuramente migliore dal punto di vista economico, continuiamo a stare vicini alle categorie più svantaggiate su questo tema. Vi è poi l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore gas e la riduzione IVA per il gas metano per combustione per usi civici e industriali. Ancora, vi è l'estensione di tali riduzioni al teleriscaldamento, che prima di questa legislatura era incomprensibilmente escluso da qualsiasi tipo di agevolazione. Vengono previste calmierazioni, con prezzi minimi e integrazione dei ricavi, per la produzione di impianti a biogas e biomasse. A riprova di un nuovo e organico approccio alla questione energetica, vi sono anche disposizioni sulla questione dell'energia geotermica, che ne prevedono l'incremento laddove opportuno. Si tratta di una fonte energetica che, con le dovute cautele, può dare un'importante contributo al piano complessivo e alla strategia sull'energia. Lo stesso discorso vale per il biometano, con le norme che consentono una procedura semplificata in caso di conversione da gas comune a biometano. Sempre in tema di semplificazioni, vanno ricordate anche le norme sulle infrastrutture strategiche in ambito energetico che vengono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili come vettori di trasporto lungo l'asse Nord-Sud e la direttrice dei dei corridoi infrastrutturali energetici europei, con conseguente priorità su tutti i procedimenti autorizzativi che le riguardano e per le proroghe motivate, che possono essere disposte anche d'ufficio. Semplificazioni a questo proposito sono presenti anche per quanto riguarda i provvedimenti espropriativi. espropriativi. Nonostante quello che alcuni incomprensibilmente dicono, analoga attenzione viene riservata anche al tema delle rinnovabili con la definizione di attività generali, in particolar modo per quelle legate all'autoconsumo svolte dal terzo settore e da imprese sociali.

quella di continuare con il sostegno - laddove necessario - rispetto al caro bollette, mentre il Governo ha lavorato e lavora alacremente, con risultati evidenti, affinché i costi energetici scendano e nello stesso tempo

che ha messo in campo una strategia energetica per la sicurezza, la prosperità e il futuro stesso della Nazione. Dopo anni di dipendenza energetica, c'è un Governo che lavora guardando all'autosufficienza come obiettivo tendenziale, assumendosi la responsabilità delle scelte, a volte anche difficili, ma mettendo le basi affinché nessuno possa decidere di chiuderci i rubinetti e metterci in ginocchio. in ginocchio. A proposito di indipendenza energetica, non ci sembrerebbe un'idea molto intelligente quella di passare dalla dipendenza dal gas russo a quella dai pannelli solari

oppositori del tema del cambiamento climatico. Certo, forse la nostra ignoranza fa sì che magari non ci scandalizziamo se a luglio fa molto caldo, e questo lo ammettiamo. non siamo certamente nostalgici del fossile, come ha detto qualcuno che, mentre stava nel Governo dei migliori, apriva le centrali a carbone, mentre il Governo Meloni, fino a prova contraria, le centrali a carbone le sta chiudendo. pertanto, andiamo avanti certamente verso la decarbonizzazione, ma con una strategia di gradualità e con la consapevolezza di non cedere alcun passo sulla sovranità in nome del politicamente corretto e dell'ideologia globalista. quindi sì alle rinnovabili. Segnalo, inoltre, ai colleghi che in questi mesi gli investimenti sulle rinnovabili che sono in campo in Italia sono ampiamente aumentati, sono triplicati rispetto a due anni fa: parliamo di 41 miliardi di investimenti sul tema delle rinnovabili e di 38 gigawatt messi in campo. mio intervento, un nuovo protagonismo dell'Italia si esplica anche sul piano Mattei, che comporta accordi non predatori con i Paesi in particolar modo del Nord Africa e sulla creazione di *partnership* plurali, tali da avere una giusta diversificazione delle fonti energetiche. Avanti così, dunque, per un'Italia che guardi al futuro e sappia coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Nella nostra visione gli esseri umani sono integrati e non contrapposti alla natura; il benessere dell'uno è direttamente proporzionale al benessere dell'altro e, visto che oggi è stato citato un proverbio dei nativi americani, ne citiamo uno anche noi: la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, ma presa in prestito dai nostri figli.

non è conviverci passivamente ma viverla in modo proattivo, non da ospiti ma da custodi. Per questi motivi, esprimiamo un convinto voto favorevole a questo provvedimento. *(Applausi)*. nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 803, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57,

chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È estratto a sorte il nome del senatore Melchiorre).*

alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Ministro, grazie per essere qui. Nel periodo estivo assistiamo costantemente a un profluvio di interviste, di servizi televisivi e giornalistici sul fenomeno dell'abbandono degli animali, un fenomeno purtroppo però non soltanto estivo, ma che concerne tutto l'arco temporale dell'anno. Nonostante migliaia di leggi emanate dal Parlamento - nella scorsa legislatura abbiamo inserito all'articolo 9 della Costituzione la tutela del benessere degli animali - siamo ancora purtroppo molto indietro nella gestione degli stessi.

Secondo «Forbes» la *pet economy* genererà 370 miliardi di dollari nel solo 2023. Eppure oggi soltanto 8,5 milioni di italiani possono andare in vacanza con il proprio animale domestico e questo perché andare in vacanza diventa un incubo.

assolutamente discrezionale. Per quanto riguarda i trasporti aerei è impensabile oggi che l'animale domestico sia considerato un bagaglio, nonostante le leggi dell'Unesco, le leggi dell'Unione europea e la nostra Costituzione, e che il cane o il gatto debbano essere messi sotto i piedi e trattati alla stregua di un trasportino e di di una valigia vera e propria. Le chiedo quindi quali misure, signor Ministro, si intendano adottare come "salva estate" nei confronti degli animali domestici e, soprattutto, dei padroni che vogliono viaggiare con loro, consentendo un'apertura che io credo sia di grande dignità e soprattutto di grande civiltà, sulla quale il nostro Paese può essere

Sul primo aspetto, relativo alla disciplina dell'accesso degli animali domestici in spiaggia, tale competenza è demandata agli enti locali e non all'autorità marittima. Visto però che il tema mi sta particolarmente a cuore, sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino misure per garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, nel rispetto ovviamente delle esigenze delle diverse tipologie di utenti. Mi farò carico, dunque, di portare il tema dell'attenzione dell'Associazione nazionale Comuni

ahimè, riconosce la legittimità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, ma non impone alcun obbligo di imbarco degli animali domestici a carico dei vettori. Anche qui, mi farò carico di l'aviazione civile (ENAC), e di sensibilizzare i vettori in merito a tale situazione. Quindi, mi attiverò con ANCI per quello che riguarda le spiagge e con ENAC per quello che riguarda il trasporto aereo. Trenitalia ospita, gratuitamente e meritoriamente, il trasporto degli animali anche in questa stagione estiva. In chiusura, grazie al suo intervento, ci è venuta un'altra idea, che penso potrà servire a dissuadere qualche incivile da un gesto di abbandono e di morte. Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale, che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando di proporre modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada e pertinenze, arrivando fino alla revoca o alla sospensione

che viaggiano. Sospensione o addirittura revoca della patente, quindi, per chi abbandona in strada un animale domestico e io spero che questo serva a far capire che dev'essere vacanza per tutti, due e quattro zampe comprese.

gli italiani che vogliono andare in vacanza e 65 milioni quelli che hanno gli animali domestici, vuol dire che c'è non solo un *gap* incredibile, ma anche una possibilità di crescita, anche economica, per il nostro Paese, che non conosce fine.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, negli ultimi dieci mesi l'Italia è stata colpita da circa 150 eventi climatici estremi, registrando danni enormi a economia, persone e territori, da Nord a Sud, da Ischia all'Emilia-Romagna. Tali eventi hanno flagellato, negli ultimi giorni, anche il Veneto e il Trentino, con effetti devastanti su agricoltura, boschi e aree naturali. Gli effetti del cambiamento climatico si stanno manifestando in tutta la loro gravità, passando da forti periodi di siccità ad alluvioni ed a temperature infuocate. Per questo motivo, è urgente intervenire con tempestività, anche a livello normativo, per mitigare gli effetti della crisi climatica in atto. Sul tema della siccità il Governo è intervenuto con un decreto-legge, convertito dalla legge n. 68 del 13 giugno 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Esso prevede, all'articolo 1, l'istituzione della cabina di regia per la crisi idrica. La stessa cabina di regia dovrebbe assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche. In data 3 maggio 2023, con il comunicato n. 784, il presidente della Regione Veneto, Zaia, ha trasmesso l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato comunicato n. 784 della Regione Veneto contiene, tra gli interventi urgenti, la realizzazione della diga di Vanoi (ad uso plurimo: acquedottistico, irriguo, idroelettrico) a Lamon, nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro. In data 4 maggio 2023, si è tenuta la prima riunione della cabina di regia per la crisi idrica, che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Considerato che il decreto siccità prevede, cito testualmente, «operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe», «individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi», «attività di esercizio e manutenzione delle dighe» e non prevede la realizzazione di nuove dighe, chiedo di sapere quale decisione intendano adottare la cabina di regia e il Governo rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi, quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo, previsto dalla richiamata legge

che mi dà l'opportunità di chiarire il lavoro fatto e di annunciare che ci sarà una seconda riunione della cabina di regia, proprio la settimana prossima, con l'audizione del commissario Parto dagli ultimi quesiti, indicando gli interventi di urgente realizzazione, per i quali il Governo ha già stanziato 102 milioni di euro, per fronteggiare la crisi idrica. Li ricordo ai colleghi e a chi ci segue da casa: in Piemonte, interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, per il risparmio idrico, del canale Regina Elena e diramatore alto novarese, per 28 milioni Lombardia, nuove opere di regolazione del lago d'Idro, in provincia di Brescia, per 33 milioni di euro; in Veneto, da lei citato, lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, di euro; in Emilia-Romagna, riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione lungo l'asta principale, opere di stabilizzazione e ripristino dell'efficienza nel tratto attenuatore-Reno del canale emiliano-romagnolo, per 13 milioni di euro; infine, nel Lazio, interconnessione per il riutilizzo dell'impianto di depurazione di Fregene, per 6 milioni di euro. Tali interventi sono stati individuati sulla base di una serie di criteri che tengono conto sia delle priorità segnalate dalle Regioni, sia delle situazioni di criticità rispetto alla risorsa idrica. È ancora in corso, ovviamente, un'attività di ricognizione per ulteriori interventi urgenti. In merito alla diga di Vanoi, da lei citata, in parallelo rispetto al lavoro della cabina di regia, il Ministero che ho l'onore di presiedere ha pubblicato un avviso per la selezione di opere nel settore idrico, il 25 ottobre 2022. Tale avviso è destinato a raccogliere e sta raccogliendo le proposte di intervento di medio periodo presentate dalle Regioni. Pertanto, il progetto per la realizzazione della diga di Vanoi potrà essere valutato dal Ministero nell'ambito di tale procedimento. Cito a memoria un'altra diga attesa da anni, che è la diga di Vetto, sull'Appennino reggiano, per la cui progettazione abbiamo stanziato 3 milioni di euro. di euro. Il lavoro sulle infrastrutture idriche, concludo, sta procedendo a ritmi serrati, nella consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di garantire al territorio gli interventi da decenni attesi. la ringrazio per la sua risposta. Purtroppo non posso ritenermi soddisfatta, anzi, sono veramente preoccupata e mi sarei aspettata che dicesse che la diga del Vanoi rimarrà nel cassetto, come lo è da quasi cent'anni,

tirare fuori dal cassetto progetti vecchi, bocciati e non sostenibili. Nel caso specifico, la diga del Vanoi ha un

si intenda procedere su questa strada, tanto più che la valle in cui dovrebbe essere inserita questa diga è stata chiusa completamente, perché è stata oggetto di una frana. Puntate su questo progetto, invece di come richiesto nel decreto-legge - a interventi di sghiaiamento per potenziare e portare a regime gli invasi (sono quattro quelli già presenti nel territorio) e senza e senza coinvolgere il territorio. Poi vi lamentate che nessuno vuole che si entri nel proprio giardino, ma dovete comunque chiedere il permesso. Lo fate senza coinvolgere

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, i Comuni, soprattutto quelli turistici, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni per violazioni al codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio provenienti dall'estero. L'articolo 196 del codice della strada prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario, quindi il turista, e non il proprietario, quindi la società di locazione, risponda in solido con l'autore della violazione. Il testo previgente dell'articolo 196, che la Corte di cassazione ha interpretato in maniera unanime nel ritenere il locatario responsabile, non lo sostituiva, ma lo aggiungeva al La *ratio* della norma era chiara: rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione. Con il decreto-legge n. 121 del 2021 si è introdotta una modifica normativa che ha escluso la responsabilità del proprietario del veicolo. La conseguenza è l'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso d'infrazione. Da qui, una perdita per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati dei locatari o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero. Tale condotta evasiva va avanti da diversi anni ed è ormai suffragata anche dalla legge, che rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio. Le chiedo pertanto, signor Ministro, se intende, in sede di esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale di sua iniziativa, prevedere una modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la *ratio* della norma sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, ormai di fatto vanificata, e introdurre ad esempio un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad avere i dati dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni ai Comuni, con la possibilità di addebito diretto degli importi sulle carte di credito prestate a garanzia del contratto di locazione, sempre che non vi sia formale contestazione del verbale di infrazione. Unterberger, intendo fare esattamente quello che lei sottolinea, perché non esiste che uno arrivi dall'estero, noleggi una macchina, prenda dieci multe in Italia e poi se ne torni a casa sua senza pagare un euro.

a noleggio senza conducente, ma tale intervento correttivo non ha consentito di superare - come mi sembra evidente - le problematiche rappresentate. Sul punto, la modifica normativa all'articolo 196 approvata nella scorsa legislatura comunque non esclude totalmente la responsabilità solidale per l'impresa locataria: soprattutto nelle locazioni di breve durata, il contenzioso è aperto. Tuttavia, quando una legge è soggetta a interpretazione, sappiamo che non è fatta bene. consapevole che sia assolutamente necessario fugare dubbi interpretativi ed evitare di onerare i Comuni di procedimenti complessi, che rendono difficoltosa l'esigibilità delle sanzioni, sono assolutamente a disposizione, anzi, auspico che questo Senato intervenga sul tema con ulteriori modifiche dell'articolo 196 del codice della strada per migliorare il disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato in Consiglio dei ministri il 27 giugno scorso e in corso di trasmissione alle Camere. Si tratta di un nuovo testo sulla sicurezza stradale che ha l'obiettivo primario di salvare vite, però vuole mettere anche un po' di ordine nella giungla del mondo delle multe, quindi normare gli autovelox a livello nazionale perché possano essere allestiti e impiantati là dove sono necessari per motivi di sicurezza, ma non servano

Presidente,signor Ministro, in questo periodo al trasporto dei pendolari per motivi di studio e di lavoro si aggiungono anche -

con un ammontare di 1.600 ore di ritardo al mese e con rimborsi talvolta non troppo definiti. A questo si aggiungono, una volta arrivati a destinazione, soprattutto nelle città turistiche, proprio per l'afflusso di turisti, le code per i taxi (che noi conosciamo); il trasporto privato vede il rincaro della benzina e anche il trasporto aereo non va meglio, con disagi, cancellazioni e purtroppo anche rincari dei biglietti, tanto che qualche settimana fa

Paghiamo una fragilità infrastrutturale causata da troppi anni senza investimenti adeguati e proprio su questo otto mesi fa, quando siamo arrivati al Governo, ci siamo messi al lavoro. Nel contratto di programma, nella parte relativa a investimenti e servizi, sottoscritto lo scorso dicembre con Rete abbiamo previsto investimenti per 23 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento tecnologico della rete e il miglioramento dei servizi. Con il PNRR sono state stanziate risorse per il potenziamento della flotta dei treni pari 800 milioni di euro. Ricordo infatti che l'Alta velocità è, sì, importante, però l'80 per cento degli italiani prende i regionali e gli *intercity.* Noi stiamo investendo miliardi di euro nell'acquisto di nuove carrozze per chi il treno non lo prende per turismo una volta ogni tanto, ma tutti i giorni per recarsi sul posto di lavoro. Per affrontare le situazioni emergenziali, ho interessato il gestore dei servizi ferroviari per disporre uno specifico piano straordinario che prevede manutenzione con precedenza alle fasce pendolari e monitoraggio della circolazione per risoluzione di eventuali criticità; c'è inoltre un piano estate, con l'attivazione di centri operativi *ad hoc*, piani di riprogrammazione dell'offerta commerciale e apertura prolungata delle stazioni. Circa i dati statistici sul ritardo dei treni, Trenitalia ha comunicato che l'indice di puntualità è passato dal 77,9 per per cento dei primi sei mesi del 2023: ovviamente questi dati, pur positivi, non bastano a soddisfarci e vogliamo ulteriormente migliorare. Quanto al trasporto aereo, l'Italia si distingue per essere tra i Paesi in cui i tagli di servizi sono contenuti, grazie ai lavoratori dei nostri scali. Proprio un'ora fa, a proposito dell'aeroporto di Catania, ho messo a disposizione, pur non essendo competenza del mio Ministero, sia della Regione sia dell'ente gestore, uomini, mezzi e, se necessario, anche attività ispettive per tornare alla normalità il prima possibile. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, ho incontrato ieri 23 sigle sindacali dei tassisti e oggi 26 sigle sindacali dei noleggi con conducente (NCC), mentre la settimana prossima ascolteremo Comuni e Regione. L'obiettivo è prima della pausa estiva, con un piano di riordino complessivo di taxi e NCC, più auto nel breve periodo e di maggiore qualità a disposizione dei cittadini italiani.

in questo racconto). Ministro, lei avrà anche convocato un tavolo, ma le ricordo che il suo è il partito che si è messo contro la riforma dei taxi in questo Paese e, se oggi c'è uno strapotere delle *lobby* dei tassisti, se non ci sono nuove licenze, se, quando si arriva a Roma si cerca un taxi, bisogna essere veramente molto fortunati a trovarlo, lo dobbiamo anche a quella scelta scellerata che è stata una delle ragioni per le quali è caduto il Governo Draghi, anche per mano vostra.

provare a percorrere anche un metro di strada per ragioni sanitarie è impossibile. E al Governo - le do una notizia - c'è lei, ministro Salvini.

*(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, con l'arrivo dell'estate aumenta l'affluenza dei turisti italiani e, per fortuna, anche di tanti stranieri nei luoghi di vacanza. Quest'anno il nostro Paese ha registrato davvero punte massime come non accadeva da tempo e soprattutto dopo la pandemia che aveva colpito pesantemente la nostra bella Penisola. Queste mete, che durante l'anno vivono un periodo di relativa tranquillità, nei mesi estivi sono chiamate a garantire maggior capacità ricettiva, oltre che di accoglienza, di organizzazione e di sicurezza per i villeggianti, perché dobbiamo consentire loro di vivere questo periodo di vacanza in totale serenità e tranquillità. Non basta quindi mostrare il biglietto da visita delle straordinarie mete e perle paesaggistiche perle paesaggistiche che caratterizzano il nostro Paese, ma è necessaria la tutela di chi viaggia per visitare anche gli angoli più remoti del nostro Paese. Ciò è ancora più importante in considerazione di quanto il turismo rappresenti un comparto importantissimo per noi e per la nostra economia. Questo non vale soltanto per i luoghi di mare e di montagna, dove ovviamente vanno garantite le operazioni di ricerca, di salvataggio e di primo soccorso, ma anche per i laghi.

un augurio per il 158° anniversario delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera italiana, che spero non vengano più tirate nella polemica politica per vicende di altro genere. *(Applausi)*. Ringrazio per l'interrogazione, che mi consente di illustrare le iniziative concrete messe in campo dal Ministero proprio in questi mesi per quello che riguarda i laghi. L'esigenza di garantire la presenza stabile della Guardia costiera sui laghi maggiori nasce dalla consapevolezza delle incrementate esigenze di mobilità lacuali. Al 30 giugno di quest'anno abbiamo infatti registrato sui grandi laghi un incremento del 22 per cento del numero di passeggeri rispetto al primo semestre del 2022. Si tratta, dall'inizio dell'anno ad oggi, di circa 5,6 milioni di passeggeri, dati che ci inducono a ritenere che quest'anno supereremo la soglia dei 10 milioni registrata l'anno scorso. Permettetemi di ringraziare anche le lavoratrici e i lavoratori della navigazione laghi, che offrono un servizio assolutamente di eccellenza. Per questo lo scorso mese di giugno, in occasione dell'avvio della campagna di sicurezza Mare sicuro 2023, ho avuto il piacere di presenziare all'inaugurazione del nuovo presidio della Guardia costiera sul lago Maggiore, finora attivo solo per i mesi estivi, e che, su mia espressa indicazione, rimarrà in pianta stabile con una sede a Lesa. Il presidio del lago di Garda è anch'esso attivo per tutto l'anno solare, con la presenza del personale della sede di Venezia. In termini di uomini e mezzi, per essere più preciso, il presidio del lago Maggiore è coperto da 16 unità della Guardia costiera e da due mezzi navali, mentre quello del lago di Garda a Salò è assicurato da 37 unità della Guardia costiera, da sette mezzi navali e da cinque mezzi terrestri. L'obiettivo a cui stiamo lavorando è quello di individuare ulteriori risorse umane e mezzi per coprire anche altri ambiti lacuali, compreso il lago di Como, mediante l'attivazione di ulteriori presidi della Guardia costiera. L'auspicio evidentemente è che questa iniziativa sul fronte della sicurezza possa essere un volano per la crescita dell'intero comparto della mobilità sugli splendidi laghi italiani. Signor Ministro, siamo noi a ringraziarla e ci riteniamo ovviamente soddisfatti per la sua risposta, perché è confortata da fatti, oltre che da numeri. Un incremento così evidente - lei appunto ha citato il 22 per cento di turisti e di passeggeri - non può che essere accompagnato da provvedimenti in grado di far fronte alle sopravvenute maggiori esigenze di copertura dei territori in termini di sicurezza. Va bene quindi anche il suo intervento per destinare più uomini e più donne della Guardia costiera a tutela dei cittadini, dei turisti e dei diportisti, che sappiamo benissimo che in questo momento sono necessari. Apprezziamo la sua sensibilità nel far fronte a esigenze di maggiore sicurezza sulla navigazione. Destinare un così importante contingente di uomini e mezzi navali, attraverso nuclei operativi ventiquattr'ore su ventiquattro, è il messaggio migliore che si possa dare a chi vuole raggiungere i grandi laghi per trascorrere un periodo di vacanza in tutta tranquillità. Ovviamente condividiamo il suo obiettivo di estendere questi presidi anche ad altri importanti bacini. Non dobbiamo dimenticare che una delle maggiori ricchezze d'Italia è rappresentata proprio dal turismo - lo dicevo in apertura - ma sarebbe un errore pensare che questo riguardi soltanto la visita delle città d'arte, caratterizzate da uno straordinario patrimonio storico, perché milioni di turisti italiani e tantissimi stranieri in in questa estate scelgono anche le zone lacustri, di collina e di montagna, per rilassarsi dopo un anno di lavoro. Lo sviluppo e la sicurezza di queste aree turistiche non potranno dunque che produrre assolutamente effetti positivi sia nel settore della mobilità lacustre, sia per quanto riguarda, come dicevamo prima, la nostra economia, che vive - e tanto - anche del comparto turistico. Quindi più sicurezza significa maggior numero di visitatori,

di tutti i siciliani e non solo, ma anche dei tanti turisti che in questi giorni hanno avuto grossissimi disagi a causa dell'incidente nell'aeroporto di Catania: grazie davvero. codice degli appalti, il rilancio degli interventi infrastrutturali e, in generale, degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale congiuntura economica, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia per una più rapida uscita dalla crisi. La ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche, nonché per la rigenerazione urbana possono assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni purtroppo si è progressivamente accentuato. Semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggior flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile e amministrativa, e soprattutto divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (il cosiddetto *gold plating*): questi sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici. L'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice ha portato a un complessivo snellimento delle procedure grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto. La revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce un obiettivo cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese. Per questo motivo, signor Ministro, essendo entrato in vigore dal 1° luglio 2023 il nuovo codice, le chiediamo se i dati disponibili in possesso del Ministero ad oggi relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano state assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti PNRR. un'accelerazione degli appalti; qualcuno pensava che si bloccasse tutto, invece il nostro obiettivo di semplificare, velocizzare e sburocratizzare, stando ai numeri che andrò a riferire, sta rendendo un buon servizio ai sindaci, alle imprese e al Paese tutto. A distanza di poche settimane dall'efficacia delle nuove regole, di cui vado orgoglioso, posso affermare che non si è registrato il rischio di uno stallo del sistema dei contratti pubblici, da qualcuno paventato. Ci sono due dati, in particolare, che testimoniano l'impegno di questo Governo a garantire che le nuove regole

aggiornati alla data di ieri, evidenziano: 5.215 istanze di qualificazione delle stazioni appaltanti presentate; 2.469 stazioni appaltanti già qualificate; 341 esonerate dalla qualificazione; solo 356 istanze respinte, pari a meno del 7 per cento in totale. Lo sfoltimento e la qualificazione delle stazioni appaltanti stanno quindi come previsto. Si tratta di un cambio di passo anche culturale per tutta la pubblica amministrazione. Il secondo dato importante riguarda i nuovi affidamenti, gli appalti, i bandi di gara - che poi sono quelli che creano

precede l'affidamento). Si tratta di un dato significativo, che testimonia che gli affidamenti stanno procedendo regolarmente e, anzi, si stanno intensificando, soprattutto se si considera che, nell'arco dell'ultima sola settimana, i CIG sono stati quasi raddoppiati, passando dai 15.471 del 12 luglio ai 29.316 del 19 luglio.

come i dati dicono - e quello che eventualmente non andrà, modificandolo. Penso però che avere un Paese più veloce, più moderno, più sicuro e con meno no e meno burocrazia sia l'obiettivo che il codice degli appalti in questi primi giorni di applicazione sta assolutamente raggiungendo. Signor Ministro, ci riteniamo pienamente soddisfatti dalla sua risposta, anche perché come Lega già dalla scorsa legislatura avevamo lavorato prima sulla delega e poi sullo schema del provvedimento, tenendo conto, come lei ha ricordato, del contributo delle associazioni,

dando maggiore fiducia a chi ce l'ha sempre chiesta (i sindaci) e sarà parte di una rivoluzione infrastrutturale, economica e sociale, che porterà sicuramente l'Italia nei prossimi anni a vivere un nuovo *boom* economico. In questo processo di sviluppo e di ripresa del nostro Paese noi saremo al suo fianco, lavorando per favorirne l'attuazione, l'attuazione, a beneficio di tutti i cittadini, di tutte le imprese, grandi, medie o piccole che siano, che sappiamo essere il pilastro dell'Italia. Grazie, signor Ministro, e buon lavoro.

Signor Presidente, signor Ministro, ai sensi della legge n. 100 del 29 giugno 2010, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia «sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia». A far tempo da marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne sottoscrivevano una nuova versione nel 2018,

protocollo n. 90, informava le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti, rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. valuta che a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica, con la conseguenza di vedere applicato ancora oggi il contratto collettivo nazionale sottoscritto il 1° giugno 2000. Considerato che i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano; considerato che, con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere pubblicistico delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari, aumentando le incertezze sulla disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti; considerato che è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria; quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore; quali azioni intenda intraprendere il Ministero della cultura, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura privatistica o pubblicistica dei rapporti di lavoro

senatore Pirondini per questo quesito, perché mi consente, innanzitutto, di aggiornare il Parlamento su ciò che il Governo e segnatamente il mio Ministero stanno facendo in questa direzione, perché stiamo profondendo molte energie su questo fronte (la vicenda viene seguita personalmente dal sottosegretario Gianmarco Mazzi). La ringrazio inoltre perché lei, sia pur implicitamente ed in maniera un po' involuta, fa un po' di autocritica, perché riconosce che il contratto è fermo da vent'anni. Allora io vi domando che cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni affinché si giungesse rapidamente ad un legittimo e sacrosanto rinnovo del contratto. *(Applausi)*. Il tema c'è, non va negato ed è legittimo e sacrosanto andare avanti. Allora io le dico, innanzitutto, che dal 2010, da quando il procedimento, non è stato fatto nulla. Noi, invece, abbiamo tenuto ben cinque tavoli con tutti gli organismi a vario titolo rappresentati, ovviamente soprattutto con le organizzazioni sindacali. L'ultimo tavolo c'è stato proprio questa mattina.

Ovviamente, ciò implica che saranno previste delle risorse, perché è evidente che non si arriva a un nuovo contratto senza una debita copertura finanziaria. Quindi, daremo le risorse adeguate affinché si possa sottoscrivere il nuovo contratto. Inoltre, mi piace ricordare, sempre a proposito del settore dello spettacolo dal vivo, che è allo studio l'elaborazione del primo codice dello spettacolo, che disciplinerà in maniera organica e moderna il settore. Sarà questa l'occasione per chiarire definitivamente la natura giuridica, pubblica o privata, del rapporto di lavoro alle dipendenze

misura attesa da anni e che il Governo si è impegnato a definire al più presto. Non appena possibile, ritengo già a breve, tale schema sarà sottoposto al Consiglio dei ministri per una approvazione preliminare.

non ha detto nulla. Il tema del rinnovo è legato alle risorse, perché è evidente che, se ci sono le risorse si fa il rinnovo, diversamente no. Sui tempi di entrata in vigore non si sa e sulla natura giuridica

sappia che noi ci siamo. Invece di fare polemiche, signor Ministro, noi facciamo delle proposte. Le chiediamo di migliorare le condizioni dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche attraverso il rinnovo del contratto delle persone che già lavorano nelle fondazioni. Le chiediamo di investire, qui sì, con orgoglio italiano, signor Ministro, in questo comparto, che da secoli dà lustro al nostro Paese. Le chiediamo di far sì che le fondazioni lirico-sinfoniche diventino uno sbocco lavorativo per i ragazzi che escono dai conservatori e che oggi hanno fondamentalmente tre opzioni: o fare i precari a vita o fare un altro mestiere oppure andare a lavorare all'estero. Quindi, è importante intervenire anche su questo. Speriamo che si possa andare nella direzione di ripristinare i corpi di danza stabili all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Su questo c'è un disegno di legge già depositato del MoVimento 5 Stelle in Commissione cultura e speriamo di poterlo portare avanti. Signor Ministro, ogni volta che non avrà voglia di fare polemica, ma voglia di risolvere i problemi, sappia che il MoVimento 5 Stelle c'è, ci sarà e farà sempre la propria parte.

signor Ministro, colleghi, voglio consegnare una premessa. Il dialogo tra le diverse articolazioni dello Stato è nel DNA del sistema territoriale dell'Emilia-Romagna, terra laboriosa, con un forte senso di appartenenza e con un orgoglio che spesso si trasforma in una preziosa responsabilità sociale. Lo hanno evidenziato i tanti volontari, ai quali vogliamo anche qui, ora, inviare un grande grazie Lo hanno evidenziato i tanti sindaci, a prescindere dal colore politico, che rappresentano insieme, credo, uno dei volti più preziosi e più importanti del Paese. una terra laboriosa, che unisce il fare al fare bene, ricercando nell'innovazione, nella ricerca, nelle trasformazioni in atto nell'economia e nella società, un'opportunità per una nuova crescita inclusiva e sostenibile. Il dialogo tra istituzioni deve rafforzarsi e non incrinarsi, essendo ancor più necessario nell'ambito di una calamità, un evento climatico senza precedenti, che ha coinvolto sette province, in un'area estremamente vasta, di 1.600 chilometri quadrati, e che, nei due eventi alluvionali, ha riversato 4 miliardi di metri cubi di acqua, quando in un intero anno, in tutta la Regione, se ne consumano 1,4 miliardi per uso civile, irriguo e industriale. Affinché il dialogo si rafforzi, signor Ministro, le chiedo innanzitutto di fermare i diversi apprendisti stregoni che spesso abitano nella sua maggioranza, in alcuni casi anche al Governo, che cercano speculazioni politiche, evidenziando responsabilità territoriali che non ci sono o negando i cambiamenti climatici, irridendo le trasformazioni ambientali in atto che, come la scienza e il mondo scientifico ci dicono, interessano l'intero pianeta. Non è razionale usare la propaganda al posto della necessaria cultura di Governo. L'intero sistema territoriale romagnolo ed emiliano, ma anche i territori colpiti della Toscana e delle Marche, non possono accettare questo declino. Signor Ministro, sono trascorsi ottanta giorni dall'inizio degli eventi alluvionali: tanti, troppi, c'è ritardo. Solo ora il generale Figliuolo, ovviamente, afferma che c'è contiguità tra emergenza e ricostruzione, l'esatto contrario di quello che il Governo aveva inizialmente sostenuto. Sempre il generale Figliuolo, che ringraziamo per il lavoro svolto, ha definito le risorse necessarie per i primi lavori di somma urgenza: sempre quei lavori che, in molti casi, lei ai nostri sindaci ha chiesto da chi erano stati autorizzati e perché li avevano avviati. Insomma, serve un cambio di passo urgente. Penso alla definizione delle risorse necessarie per indennizzare famiglie e imprese al 100 per cento, come promesso dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni *(Applausi)*. Lavoriamo ogni giorno per smentire le sue previsioni, dichiarazioni fuori tempo e fuori dal tempo, secondo le quali servono nove anni per la ricostruzione. Speriamo di trovare nel suo Governo un alleato. Servono rapidità ed efficienza, servono misure straordinarie e regole semplici. Abbiamo bisogno di ricostruire in fretta il bacino idrografico, per mettere questo territorio in sicurezza e per garantire all'intero Paese la produzione lorda vendibile, che nel settore agricolo è così fondamentale. Servono risorse urgenti anche per il comparto dell'agricoltura. Ancora non abbiamo un quadro economico chiaro e preciso, finalizzato a salvaguardare la credibilità del suo Governo e dunque la credibilità di tutte le istituzioni. Fate in fretta, perché in gioco c'è la democrazia e soprattutto ci sono la fiducia e l'affidabilità, che devono essere garantite a questo sistema territoriale, che ha sempre garantito all'intero Paese, non solo la locomotiva dello sviluppo economico, ma anche un luogo fondamentale di partecipazione e di vita democratica.

Onorevole senatore, aderendo al suo invito, mi attengo a un profilo istituzionale assolutamente governativo e mi permetta di dirle che non raccolgo la sua polemica,

confidando nella clemenza della Presidenza se abuserò di qualche secondo in più. Per quanto riguarda le aperture dei cantieri dei sindaci, il sottoscritto non ha mai messo in discussione, né può perché lo prevede la legge, il diritto dei sindaci ad aprire cantieri di iniziativa, nel regime emergenziale, perché lo prevede il codice di protezione civile. Il riferimento era per la fase della ricostruzione, perché, come lei sa e come sanno gli onorevoli senatori, non esiste una norma che definisca con assoluta chiarezza - in questo senso stiamo provvedendo - dove finisce lo stato di emergenza e dove inizia quello della ricostruzione. Quanto ai nove anni, pensavo che la proiezione del video del mio intervento fosse sufficiente, ma naturalmente mi rendo conto che non è bastato. Questa è l'occasione propizia per riproporre il tema: in Italia non esiste una norma che preveda quanto debba durare lo stato di ricostruzione. Nella valle del Belice dal 1968 è ancora incompleta, lo stesso in Irpinia,

a tutte le fasi di ricostruzione. Tutte significa alluvione, significa dissesto, significa incendi, significa crisi industriale, significa sisma; il termine massimo che noi prevediamo è di dieci anni per qualunque tipo di ricostruzione. *(Applausi)*. È chiaro che una cosa è ricostruire un territorio dopo un'alluvione,

che avrebbe dovuto allarmare le opposizioni, visto che in Italia le ricostruzioni possono durare anche quarant'anni, ma invece di raccogliere consenso mi è sembrato un argomento per una polemica davvero di cattivo gusto. Tuttavia, se mi consente, torno al testo: Manca, che dopo i primi provvedimenti di carattere strettamente emergenziale, il Consiglio dei ministri ha approvato un primo decreto-legge per garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e quindi procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. Mi scuso per la rapida lettura, per non abusare del tempo concessomi dalla Presidenza: con successivo decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, sono stati definiti i principi organizzativi e le misure normative per assicurare un pronto avvio della ricostruzione, sia pubblica che privata. Il decreto di ricostruzione è stato trasfuso nel decreto alluvioni, con emendamento approvato dall'VIII Commissione della Camera nella seduta di ieri. Quest'ultimo provvedimento, con cui è stato pure istituito un apposito fondo per la ricostruzione, che non è mai esistito in Italia dal dopoguerra ad oggi *(Applausi)* (questa è una responsabilità, se mi consente, *bipartisan*, di tutti gli schieramenti), ha istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro per il triennio 2023-2025 e contiene, tra l'altro, specifiche misure per la pianificazione degli interventi su situazioni di dissesto idrogeologico e per la ricostruzione delle infrastrutture ambientali danneggiate. Si tratta di misure che si aggiungono a quelle già previste da altre disposizioni straordinarie, prima fra tutte quelle istitutive della gestione commissariale deputata al contrasto del dissesto. Il provvedimento consente inoltre di velocizzare le procedure di ricostruzione, sia mediante specifiche deroghe normative, sia attraverso l'attribuzione del potere di ordinanza al commissario straordinario per la ricostruzione. Il commissario è competente a disciplinare in deroga, anche introducendo le occorrenti misure di semplificazione, e a erogare in via diretta i contributi per la ricostruzione privata fino al 100 per cento delle spese occorrenti e nei limiti naturalmente delle disponibilità esistenti. Sono previste anche specifiche misure di sostegno in favore delle famiglie dell'Emilia-Romagna. In particolare, è stato autorizzato un contributo entro il limite di 5.000 euro finalizzato al ripristino dei danni all'abitazione, agli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, alla sostituzione o di beni mobili distrutti o danneggiati. A quello appena citato può aggiungersi un contributo forfettario di 750 euro per il concorso alle spese di perizia e uno, sempre per un massimo di 5.000 euro, per il ripristino delle parti comuni degli edifici condominiali non fruibili. Tali misure, che costituiscono un immediato sostegno ai privati, hanno visto finora circa 17.000 domande presentate; alla data del 16 luglio scorso sono stati erogati i primi 2.700 acconti ed entro il 23 luglio

Signora Presidente,ovviamente non siamo affatto soddisfatti, per due ragioni fondamentali. In primo luogo, noi riconosciamo la legittimità della scelta del Governo di non utilizzare strutture commissariali già presenti in Emilia Romagna; avete scelto una strada, quella di costruire una struttura nazionale con un commissario, alternativa all'utilizzo di una struttura. Questo è legittimo, però non accettiamo che lei racconti cose non vere sulla ricostruzione post terremoto perché ci sono le parole di tanti Governi, quelle del Presidente della Repubblica, quelle di tanti suoi colleghi che hanno visto come la ricostruzione è stata possibile, perché è stata perché immediatamente i Governi di allora hanno deciso che venissero ricostruite le case delle persone riconoscendo il 100 per cento dei danni. Tutto ciò da subito. Non sono trascorsi giorni: dopo otto giorni le regole fondamentali della ricostruzione erano definite. In questo caso sono trascorsi ottanta giorni e non c'è un quadro economico e finanziario che rispetta le promesse che il Governo ha fatto in quel territorio. Non ci impedirete, nella lealtà e nella leale collaborazione, di richiamare il Governo ogni giorno alle proprie responsabilità. Questo è il senso del nostro intervento; anzi, le diciamo con grande chiarezza che se aveste definito la cornice economica e finanziaria, anche con uno scostamento dagli obiettivi di medio termine, noi lo avremmo votato e sostenuto. Invece ancora oggi le risorse per indennizzare le famiglie e le imprese e per mettere in sicurezza quel territorio non ci sono. Noi vi chiameremo alle vostre responsabilità. La ricostruzione del terremoto è stata virtuosa, utile e importante anche per riconsegnare al Paese una crescita economica di quelle aree superiore a quella che c'era prima del terremoto. prima del terremoto. Questo è l'elemento che più di tutti ci distingue e ci distanzia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in quel territorio; chiediamo al Governo di fare la stessa cosa, se ci riesce, con le scelte politiche che noi non che noi non condividiamo, ma che sono legittime, che ha sviluppato in questi mesi, durante i quali a mio avviso si è perso troppo tempo e si sono fatte più passerelle che fatti.

tutela del territorio, a una mancata pulizia degli argini che più volte era stata denunciata anche dal sottoscritto all'epoca in Consiglio regionale e a cui purtroppo non era stata data risposta né dal presidente Bonaccini, né dall'allora assessore ai cambiamenti climatici Elly Schlein.

Il Governo ha messo in campo subito quattro provvedimenti, dai primi decreti di maggio fino a quelli di luglio, che hanno inizialmente stanziato 30 milioni per le somme urgenze, cosa che non era mai accaduta in in passato, quindi oltre 4 miliardi con i decreti, con la struttura commissariale che grazie al cielo è gestita dal generale Figliuolo, perché oggettivamente sentir

realtà mancavano alcuni Comuni che però hanno avuto dei danni derivanti dall'alluvione, nonostante lo stato di emergenza riguardasse appunto le Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

Onorevole senatore, lei ha fatto riferimento alla struttura per la ricostruzione *post*-sisma. In effetti, la struttura è ancora in vita, perché si deve completare la procedura di definizione, come ho detto poco fa, molta parte dei lavori, dopo undici anni, risulta essere stata realizzata, il che mi conforta nel senso che il termine massimo per le ricostruzioni da calamità di dieci anni credo possa essere ragionevolmente accettato. Il quadro economico-finanziario della ricostruzione in Emilia-Romagna è competenza del commissario straordinario, non è competenza del Governo e penso che il commissario dovrà e potrà provvedere nei prossimi giorni, d'intesa con il Presidente della Regione che abbiamo designato come subcommissario, e naturalmente degli enti locali. Lei e tutti i colleghi ricorderete che il Consiglio dei ministri, con delibera del 4 maggio, ha istituito per dodici mesi lo stato di emergenza in relazione alle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, stanziando 10 milioni di euro, ma lo ha ricordato lei e non mi soffermo su questo concetto. Quello che a me piace ricordare è invece che è necessario evidenziare, in risposta al suo quesito, come sia le attività di protezione civile, sia quelle di ricostruzione riguardino l'intero territorio colpito dagli eventi alluvionali per cui sono stati riscontrati i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza. Con particolare riguardo all'Emilia-Romagna, le delibere del Consiglio dei ministri del 4 e del 23 maggio fanno riferimento alle Province di cui ho appena parlato e si tratta quindi di una perimetrazione che non si basa su ambiti comunali, ma su aree provinciali, pertanto le misure di sicurezza e assistenza alla popolazione tipiche del regime di protezione civile, sono attuate in relazione a tutti i Comuni delle Province indicate, senza che rilevi in senso limitativo l'elenco di cui all'allegato 1. Lo stesso decreto-legge alluvioni richiama l'allegato 1 soltanto in alcune specifiche disposizioni e non certamente per l'applicazione di altri provvedimenti e provvidenze in cui si fa riferimento all'ambito territoriale in stato di emergenza. Per quanto riguarda le misure del decreto-legge n. 88, oggi trasfuso nel decreto-legge alluvioni, l'ambito di applicazione non riguarda solo i territori dell'allegato 1, essendo possibile l'azione commissariale di ricostruzione anche per quei territori che, pur non indicati nell'allegato, sono stati danneggiati dall'alluvione e sono dunque compresi nelle delibere di stato di emergenza. A tali fini occorre la dimostrazione, con una perizia asseverata, che il danneggiamento è collegato agli eventi alluvionali, per evitare una ricostruzione slegata dalla calamità. In ogni caso, ho il piacere di riferire che nella giornata di ieri l'VIII Commissione della Camera ha approvato un apposito emendamento, riformulato su iniziativa del Governo, che ha assegnato al commissario straordinario il compito di provvedere, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni nei quali si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso.

di fatto ha avuto diversi danni dalle frane, ma i cui Comuni non rientravano in quell'allegato. Quindi è con soddisfazione che noto che il Governo ancora una volta va a riempire le lacune rispetto alla segnalazione che aveva fatto la Regione Emilia-Romagna. Dopodiché io mi permetto, anche rispetto alla sua conclusione, di segnalarle pubblicamente una cosa, che comunicherò anche al generare Figliuolo, ovvero alcune richieste di danni che ci lasciano parecchio perplessi, rispetto ad alcuni Comuni che hanno inserito immobili già danneggiati, ma che non sono stati danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio, i quali evidentemente rientrano però nelle richieste che vengono fatte. fatte. Se da un lato è assolutamente necessario, al contrario di quello che è avvenuto per l'alluvione del 2014 a Bomporto e a Bastiglia e al contrario di quello che avvenuto due anni e mezzo fa a Nonantola, un rimborso al 100 per cento integrale per tutti coloro i quali hanno perso qualcosa,

che se ne è approfittato per far sì che aumentassero gli sprechi. Così non deve essere; abbiamo fiducia sia nel Governo che nella nuova struttura commissariale, per il bene degli emiliano-romagnoli.